L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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 Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi»

che siamo di fronte a una vera e propria strage che continua in tutti i settori, comparti, dimensioni di azienda, realtà private o contesti pubblici. Nessuno può dirsi esente dal problema del rischio che troppo spesso è ricorrente. Per questa ragione ritengo che continuare a insistere solo sul fronte delle politiche legislative e delle norme non sia efficace e non ci protegga da questi rischi.

riferimento alla formazione, alla responsabilità, eccetera. Se una ditta appalta e subappalta deve sapere che è responsabile della filiera della produzione e non si può saltare questo tipo di ragionamento, perché sennò continuiamo a piangere

che bisogna fare un ragionamento solo di tipo sanzionatorio. Da qui l'idea - che mi pare importante - di costruire una *governance*, perché questo è l'altro dato fondamentale. Bisogna mettere insieme gli enti, e trovare un luogo in cui questi soggetti si parlano, costruiscono e intervengono collettivamente e in modo coordinato.

ho convocato per il prossimo giovedì mattina l'Ufficio di Presidenza della Commissione d'inchiesta che avrà il compito di affrontare questo tema, sottolineando che il nostro compito non è quello di interferire con quello che la magistratura ordinaria dovrà fare. Il nostro compito è capire

La invito a terminare.

Signor Presidente, il senatore Magni ha detto praticamente tutto quello che c'era da dire, ma io vorrei integrare con una considerazione legata alla mia storia personale. Ho cominciato a lavorare anni fa per pagarmi gli studi e ricordo perfettamente allora com'erano i cantieri edili, come si lavorava sulle strade. Eravamo in condizioni assolutamente libere, non c'era praticamente nessuna forma di prevenzione rispetto agli infortuni sul lavoro, se non la buona volontà dei datori di lavoro di allora o dei committenti. Se n'è fatta di strada da allora e abbiamo adesso un sistema che non possiamo buttare a mare soltanto perché succedono continuamente episodi come questi. Dobbiamo piuttosto valorizzare le norme che ci siamo dati e i modi che i modi che il nostro Paese si è dato per garantire la sicurezza sul lavoro, perché evidentemente c'è qualche passaggio che non funziona. Affinché questo sia possibile, non ha senso, colleghe e colleghi, Presidente, pretendere di pretendere di fare proposte di parte. Mettiamoci tutti insieme; il Paese adesso si aspetta che l'organo legislativo, il Senato, ma anche la Camera, si mettano insieme e propongano qualcosa che risolva il problema. Come dice il senatore Magni, lavoriamoci insieme, ma davvero questa volta, perché è un tema che non può diventare di qualcuno, ma dev'essere di tutti, a favore del nostro futuro. *(Applausi)*.

che sia un atto dovuto e doveroso da parte di quest'Assemblea riflettere con grande attenzione sui drammatici fatti di Firenze. Nell'esprimere cordoglio e solidarietà ai familiari e alla comunità colpiti, non possiamo però non esimerci da qualche riflessione più puntuale e più profonda, sia pure contingentata nei tempi e nei termini in cui la nostra discussione si deve svolgere. Infatti, se vogliamo evitare che questo si trasformi in una dinamica di ritualità, in cui la retorica tende sostanzialmente ad attutire, quando non ad annullare, gli elementi che spettano alla politica in termini di capacità di intervento e di prevenzione, non possiamo non considerare che vi sono o vi possono e vi devono essere una serie di interventi che la politica, le istituzioni e il legislatore debbono compiere sotto questo versante. Devono essere fatte anche delle assunzioni di responsabilità che considerino con grande attenzione anche alcune scelte che sono state compiute, sia in ordine alla modifica di alcuni aspetti legislativi (penso alla modifica del codice degli appalti, con l'introduzione della possibilità di una serie di subappalti a catena, che sostanzialmente vanno nella direzione di una dequalificazione del sistema delle imprese, che comporta quindi il fatto che i costi vadano a scapito della qualità, della tutela e della possibilità di garantire forza lavoro formata e

manichea nella quale troppo spesso ci infiliamo, per considerare in maniera oggettiva e il più possibile relativa gli elementi che ci impongono di fare i conti con i dati che ci sono stati forniti, che sono assolutamente inaccettabili dal punto di vista numerico e della modalità con la quale nel nostro Paese abbiamo dei caduti sul posto di lavoro (perché così li dobbiamo definire), tutto questo non può che imporci - al di là, lo ribadisco, di una necessaria, indispensabile ed esigente attività di ricordo - anche una capacità di valutazioni prospettiche. Mi faccia dire, signor Presidente, in conclusione, che l'elemento che sembra emergere da questi fatti - che cioè in quel contesto vi fossero anche anche immigrati irregolari - non può che farci interrogare ulteriormente circa il fatto che si sta chiudendo, in maniera quasi beffarda, la conseguenza di una nostra incapacità di governare un fenomeno che poi, in maniera

alle famiglie delle vittime. Nella mia vita non parlamentare sono stato a mia volta responsabile di cantieri legati all'edilizia per tanti anni e so di cosa si sta parlando. Quando ho visto la tragedia di Firenze, ho pensato a quattro grandi tragedie che sono capitate sul mio territorio, il Piemonte: la gru in via Genova, crollata con tre morti; la tragedia della ThyssenKrupp; la tragedia dell'amianto dell'Eternit; la strage ferroviaria di Brandizzo.

Probabilmente dobbiamo investire di più sulla cultura della sicurezza, sulla formazione alla sicurezza, sulla formazione al rispetto delle regole, perché la tragedia di Firenze ha qualcosa di incomprensibile, posto che si trattava di un cantiere molto grande, dove non solo le norme di sicurezza sono di un livello più elevato, ma dove anche l'organizzazione del lavoro dovrebbe portare a razionalizzare gli interventi sulle strutture. per prima cosa si dovrebbe avere un controllo più puntuale sulle fasi di lavoro nelle diverse aree del cantiere. Sarebbe gravissimo se una squadra fosse intervenuta per proseguire con un lavoro senza essere a conoscenza del fatto che il lavoro di fissaggio di una trave non era terminato. giusto quindi invocare controlli esterni, ma il primo controllo deve essere interno. Devono essere rispettate le regole, così come vogliono anche gli imprenditori seri. La prima regola da osservare è il rispetto rigoroso delle regole. Su questo tema abbiamo anche presentato, proprio in questi giorni, una proposta di legge a prima firma della senatrice Ternullo, per istituire la patente a punti sulla sicurezza nei cantieri ad alto rischio. Dobbiamo ancora lavorare per arrivare a far sì che ogni lavoratore, ogni giorno, possa lavorare in sicurezza e tornare in salute dai suoi cari. Continuiamo a impegnarci per questa che sembra un'ovvietà, ma la dobbiamo purtroppo ancora trasformare in realtà. Signor Presidente, anche noi ci associamo alle parole dei colleghi che ci hanno preceduto. Sui temi relativi alla sicurezza sul lavoro e alle morti sul lavoro troppe volte ci siamo trovati in quest'Aula commemorare e dire più o meno le stesse cose che stiamo ripetendo oggi. Sicuramente ci sono stati dei passi avanti; abbiamo letto anche noi le dichiarazioni della ministra Calderone. Ci troviamo sicuramente d'accordo con di insegnare la sicurezza sul lavoro a tutti i livelli, a partire già dalle scuole, proposta che, tra l'altro, anche noi avevamo avanzato diverse volte. Sicuramente il sistema degli appalti e dei subappalti a cascata non favorisce l'applicazione delle norme che pure esistono, quindi una riflessione su questi sistemi va certamente fatta e le modifiche recenti probabilmente andrebbero rettificate e riportate a un sistema più limitato e più suscettibile di essere verificato e controllato come si deve, per evitare che incidenti come questi possano accadere di nuovo. Infatti, come diceva il senatore Rosso, se manca la comunicazione e il dialogo, sicuramente avviene perché le strutture sono indipendenti e non dialogano tra di loro. Se questo fosse limitato, ci sarebbero più tutele per i lavoratori che sono l'ultima maglia della catena, l'ultimo anello e quelli che ne pagano le conseguenze peggiori. Noi ribadiamo, come abbiamo fatto già altre volte, la speranza che finalmente tutti insieme ci si renda conto della necessità di una procura nazionale del lavoro che riesca a congiungere in sé tutte le competenze e le specificità su questi temi cruciali per la vita dei lavoratori, perché parliamo proprio di vita in senso stretto. Ci auguriamo quindi che si possa giungere anche a questa realizzazione, insieme a tutte le altre, di comune accordo, perché penso che l'intento comune sia quello di garantire che chi esce la mattina di casa per andare a lavorare torni a casa la sera in salute. Signor presidente Centinaio, le rivolgo la nostra solidarietà per la minaccia anonima che l'ha raggiunta al proprio domicilio. Sappia che ha vicino la Lega e credo anche tutti gli altri colleghi di questa assise. *(Applausi)*. Il tempo è poco e devo purtroppo intervenire su una tragedia che ha colpito, nella mia Toscana, la città di Firenze. Una tragedia che purtroppo ha palesato gravi criticità nella fase di formazione tecnica e di sorveglianza all'interno dei cantieri. Questo nel momento in cui il mercato è spinto in maniera veramente virulenta dall'incentivo che l'edilizia ha trovato, dapprima sui *bonus* edilizi e poi sugli ingenti fondi PNRR, che evidentemente hanno totalmente assorbito la manodopera disponibile per proseguire con le tante opere aperte. Si è palesata, evidentemente, in questo cantiere una grave serie di inadempienze o di sottovalutazioni, ma sarà la magistratura, che molto diligentemente si è posta al lavoro, silenziosamente, a chiarire cosa è accaduto. Mi sia permesso rispondere a chi, in questi giorni, ha voluto criminalizzare la generalità dei subappaltatori: meno male che esistono, perché altrimenti questo Paese non avrebbe potuto dare corso ai tantissimi cantieri che, grazie ai fondi PNRR, stanno modernizzando il Paese. Secondo punto, non è assolutamente corretto andare verso un ulteriore inasprimento della normativa criminale. Qualcuno ha detto che non si può morire per mille euro al mese. Io chiedo, allora, se è giusto morire per 2.500 euro o se è giusto morire per 3.000 euro? Non è mai giusto morire, figuriamoci per una qualunque somma, che non può quantificare il dolore delle famiglie. Se qui c'è qualcosa da fare, è incentivare le aziende a monitorare costantemente i cantieri, anche utilizzando le moderne tecnologie di ripresa

di regolazione degli ingressi in Italia dei lavoratori stranieri, ha imposto e premiato quei lavoratori che possono completare in patria corsi di formazione e anche il possesso, ovviamente, dei requisiti linguistici. Siamo vicini alle famiglie, ci stringiamo al loro dolore e che mai più queste tragedie accadano, in Italia e neanche in altri posti del mondo.

rispetto al misurarsi con una strage sul lavoro. Non è la prima volta che lo facciamo in questa legislatura e non è certamente la prima volta che lo facciamo in quest'Aula, negli anni che abbiamo alle spalle. tendiamo a versare lacrime di coccodrillo, perché poi, alcuni giorni dopo, l'argomento cade nel dimenticatoio e si aspetta il successivo avvenimento. Io credo che, davvero, l'impegno che potremmo prendere, essendo noi l'Aula

escono dalla retorica che troppo spesso ha caratterizzato questa discussione: i costi, i vincoli, il non poter pretendere. Noi dobbiamo dire che si può pretendere che non si muoia sul lavoro. Si può pretendere che quei mille morti all'anno, che sono una soglia da cui non riusciamo a scendere, diventino Il caso in questione, che non è tanto diverso da quello, ahimè, avvenuto a Brandizzo, ci dice delle cose precise. In questo Paese mancano i controlli. Bisogna assumere gli ispettori e bisogna farli lavorare. E bisogna farli lavorare nelle condizioni migliori. Non possono esserci preavvisi e annunci: forse verrò e, nel caso, in che giorno preferite? No, devono esserci i controlli, come vale per tante altre E non è vero che è sempre meglio l'incentivo. Qualche volta è meglio la sanzione. Il secondo punto su cui bisogna ragionare è quale sia la responsabilità dei committenti. Noi abbiamo, come sistema pubblico, giustamente, una responsabilità dei committenti e non si capisce perché nel sistema privato non possa essere lo stesso. Perché non ci sia quella norma che impone, a chi concede degli appalti, non solo di verificare la regolarità delle retribuzioni e delle regolarità contributive, ma imponga anche di verificare l'applicazione del corretto contratto e delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Usare un contratto che non è quello giusto, infatti, innanzitutto mette in condizione di insicurezza i lavoratori e li espone a dei pericoli. Non serve una grande, nuova legislazione. Ce l'abbiamo e, per molti aspetti, funziona anche. Non funziona quando non la si controlla e quando non la si rende cogente nel sistema degli appalti. Io credo che se riuscissimo a impegnarci su queste due cose potremmo raggiungere quello che credo che sia un obiettivo condiviso, che i morti sul lavoro diminuiscano e non siano più - ahimè - l'oggetto quotidiano delle notizie, perché non dimentichiamoci che noi parliamo nei giorni delle stragi, ma ogni giorno muore qualcuno sul lavoro e quel qualcuno ha lo stesso diritto di tutti gli altri di poter tornare a casa, invece che perdere la vita.

hanno comportato, sia per il modo in cui è avvenuto questo grave infortunio mortale. Il silenzio davanti all'accaduto appare quindi inizialmente la forma più rispettosa per manifestare il cordoglio, il rispetto, per essere vicini a tutti coloro che stanno soffrendo: le famiglie, gli amici, i colleghi (non dimentichiamoci dei colleghi). Un silenzio rispettoso del dolore, ma anche denso di partecipazione, quella partecipazione che da subito questo Governo non ha mancato. Il tempo del silenzio lascia però subito l'iniziativa a un'immediata, a una necessaria, a una forte responsabilità. Oggi è veramente il tempo della responsabilità. Oggi non occorrono più proclami - l'abbiamo detto tutti - non servono più solo parole o sterili polemiche, come si sono sentite in queste ore (è inutile negarlo). Occorre la correttezza e la concretezza del fare. Insieme al mondo delle imprese, insieme agli istituti che vi sono preposti e insieme alle rappresentanze dei lavoratori occorre porre e poi mantenere la cultura della sicurezza. Oggi abbiamo una sola parola d'ordine: prevenzione. Questa si traduce in una delimitazione dei rischi, in una corretta informazione, in percorsi di formazione di cui tutti spesso parliamo, ma che dobbiamo sempre più concretizzare. Al tempo stesso, sono convinta sia necessario introdurre maggiori controlli (lo siamo tutti noi), ma controlli mirati. È necessario iniziare da lì, con il supporto di una stretta normativa e - perché no? - se sarà necessario, senza escludere la possibilità di introdurre il reato di omicidio Non credo che siamo stati con le mani in mano in questo primo periodo. Tutti - e dico tutti - ci siamo dati da fare. Il mondo del lavoro e tutti i suoi attori protagonisti aspettano delle risposte:

già ieri lo ha fatto il nostro capogruppo Boccia, in dichiarazioni pubbliche. Ma anche in questa sede, soprattutto vedendo la sua Presidenza, vorrei intervenire per esprimere a lei la nostra vicinanza e la nostra solidarietà per il grave atto di intimidazione

la magistratura faccia subito piena luce), siamo certi che né lei, naturalmente, né nessuno delle istituzioni si lascerà intimidire da chiunque voglia usare questi metodi, che non fanno ovviamente parte del confronto politico, ma neppure di una minima convivenza civile.

Comporta intanto una maggiore incisività e convinzione che si sta agendo nel giusto e sono certo che questo è il sentimento che la accompagna e che continuerà ad accompagnarla nella sua attività politica. Si tratta, però, certamente di un atto molto spiacevole da subire e per questo esprimo la nostra più grande e sentita vicinanza.

particolarmente incisive perché proprio a casa sua, e questo indica anche una

Signor Presidente, approfitto della circostanza per manifestare anche pubblicamente le considerazioni che ho già avuto modo di farle in forma privata. Tuttavia, avendo i colleghi giustamente introdotto una discussione di questa natura, nel manifestare la solidarietà del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe a lei, signor Presidente, vorrei dire che chi minaccia il Vice Presidente del Senato, chiunque esso sia, minaccia la democrazia di un Paese e minaccia il Parlamento, che rappresenta i cittadini. *(Applausi)*. Dobbiamo quindi manifestare tutti un sentimento di umana solidarietà nei confronti suoi e della sua famiglia. Ma dobbiamo dire con grande nettezza e chiarezza che questi gesti sono inaccettabili perché colpiscono i simboli su cui si regge l'impalcatura della nostra democrazia rappresentativa. Questo vale per quanto accaduto nei confronti del vice presidente Centinaio, ma anche - lo voglio dire al presidente Malan, perché ho già avuto modo di dirlo pubblicamente - nei confronti della inaccettabile scena che è accaduta sabato a Torino, quando, all'interno di una manifestazione pubblica, alcuni facinorosi hanno ben pensato di bruciare le fotografie della Presidente del Consiglio e del presidente Netanyahu. Quando noi non siamo d'accordo con la presidente del Consiglio Meloni o col presidente Netanyahu, facciamo quello che la democrazia esige e prevede: veniamo in quest'Aula e lo diciamo *(Applausi)*. Ma, quando si passa dalle parole alle vie di fatto e quando si confondono la tutela e il diritto delle persone, che sono sacri, con la manifestazione delle proprie idee, pensando che le persone possano essere sottoposte a violenze, quella non è più democrazia, ma è un'altra cosa che noi condanniamo in maniera assoluta. Signor Presidente, anche il Gruppo per le Autonomie si associa all'espressione di solidarietà nei suoi confronti per i fatti accaduti. Ormai chi mi ha preceduto quasi tutto. Rimane solo da confermare che la libertà di esprimere il proprio pensiero e di svolgere attività politica in maniera corretta, che l'ha sempre contraddistinta anche nel contraddittorio politico, merita veramente apprezzamento e vicinanza particolare. particolare. Le idee vanno sempre difese. Inoltre la libertà di esercizio del pensiero politico è un valore troppo grande perché possa essere compromesso da minacce di qualunque tipo. Siamo dunque certi che le minacce non faranno sicuramente modificare i comportamenti, ma è importante anche sentire la solidarietà dei colleghi che operano in Senato.

un conto sono la lotta politica, le opinioni e le idee, un altro conto è utilizzare strumenti che non ci appartengono e non possono appartenere a un dibattito e a un confronto civili.

Presidente, anche il Gruppo Forza Italia si associa alle parole di solidarietà e sostegno alla sua figura che sono state pronunciate da diversi esponenti in quest'Aula. L'atto intimidatorio di cui lei è stato vittima è particolarmente vile e va condannato in modo netto. La battaglia politica può avere anche degli scontri e dei toni accesi, ma non deve mai sfociare in violenza: questo fa parte delle regole della democrazia e credo che vada riaffermato oggi, una volta di più, evitando di tornare a tragiche pagine del passato che hanno insanguinato la storia di questo Paese. Quindi, ribadiamo la nostra massima solidarietà a sostegno e siamo sicuri che questi vili atti intimidatori non saranno in grado di condizionare il suo operato sia come Vice Presidente del Senato, sia per quanto riguarda la sua attività politica, che sicuramente è cristallina e lineare nella sua azione. *(Applausi)*.

all'amico Gian Marco Centinaio, nonché Vice Presidente del Senato. Questo mio intervento è rivolto soprattutto agli altri colleghi di tutti i partiti, che ringrazio per l'intervento e la solidarietà espressa. Questo può essere un principio anche di un segnale che vuole anche un po' cambiare un clima che purtroppo si vede a livello politico e culturale nel nostro Paese; cui si vedono più odio, livore e astio in qualsiasi tipo di intervento. Ci sono troppi insulti, anche da parte di persone che ricoprono importanti ruoli istituzionali e che dovrebbero dare l'esempio. contestazioni e l'impossibilità di poter esprimere determinate idee in situazioni che una democrazia dovrebbe consentire invece di poter fare. La politica può e deve dare l'esempio. Quindi, oggi è una giornata importante, in cui raccogliamo

anche tra di noi tante volte. Qualcuno dice che faccio troppo il democristiano quando dico queste cose, ma in realtà è un invito alla mitezza, nel senso che ci si può confrontare anche duramente, anche portando avanti le proprie idee con passione e determinazione, ma sempre

di più e anche la nostra democrazia, la nostra libera espressione, il fare politica e il ruolo della politica rischiano di diventare sempre più difficili, sempre più complicati. Si rischia

e vicinanza all'amico Gian Marco Centinaio. ricevere un proiettile a casa nella propria casella della posta è devastante dal punto di vista personale, ma soprattutto dal punto di vista familiare. Vi ringrazio quindi non solamente come Gian Marco Centinaio e come Vice Presidente del Senato o persona che fa politica, ma anche a nome della mia famiglia, perché sono state ore abbastanza importanti. *(Appalusi)*. Lo dico molto onestamente.

di cui agli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il relatore, senatore Salvitti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-*ter* e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto superbonus per le quali, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2003, è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. Il comma 2 riconosce inoltre ai cittadini con reddito di riferimento non superiore ai 15.000 euro, che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento entro il 31 dicembre 2023, uno specifico contributo. L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta attraverso la cessione del credito e dello sconto in fattura dell'agevolazione fiscale anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici alle zone sismiche 1, 2 e 3 comprese in piani di recupero di patrimonio patrimonio edilizio o riqualificazione urbana per le quali non sia stato richiesto prima del 30 dicembre 2023 il relativo titolo abilitativo. Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscano della detrazione al 110 per cento (superbonus) per interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici. L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del decreto-legge n. 34 del 2020. Le norme in esame restringono dal 30 dicembre 2023 l'ambito oggettivo dell'agevolazione. Essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che, per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti debbano essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il corrispettivo dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolativi di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche in alcune specifiche ipotesi. Inoltre lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023 risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo, ove necessario, ove non sia prevista, ove siano iniziati i lavori oppure nel caso in cui lavori non siano ancora iniziati e sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

siamo impegnati nella discussione generale di uno dei provvedimenti più controversi e politicamente rilevanti dall'avvio della legislatura. È una misura, quella del superbonus, che coinvolge allo stesso tempo le politiche energetiche, le politiche fiscali, gli incentivi all'occupazione, il sostegno allo sviluppo e la transizione ecologica del Paese, oltre alla vita di famiglie e imprese. È un provvedimento che riguarda i *bonus* edilizi, ma, che rispetto alle valutazioni e alle conseguenti determinazioni che sta compiendo il Governo, svela le linee di indirizzo che animano la maggioranza e le forze politiche che la sostengono. Prima di entrare nel merito delle questioni di dettaglio, dobbiamo assumere come presupposto imprescindibile una premessa, un punto di chiarezza che ci possa accompagnare con cognizione di causa nel corso di tutta la nostra discussione e poi, nei mesi a seguire, sul dibattito che non si fermerà al voto di oggi. Dobbiamo dire, con chiarezza e senza tema di smentita, che sulla vicenda del superbonus da parte del Governo è stata messa in campo la più grande operazione di propaganda degli ultimi decenni; una narrazione demolitoria verso questa misura, dapprima propagandata per ragioni ideologiche ed elettorali contro le forze politiche e i Governi che l'hanno sostenuta; poi via via evoluta in una narrazione giustificatoria, in un alibi, in sostanza, che ha trasformato i *bonus* edilizi nell'origine di tutti i mali per la finanza pubblica e, dunque, per giustificare una manovra finanziaria assolutamente inadeguata. la Presidente del Consiglio, dopo svariati improvvidi interventi sul tema di autorevoli esponenti del Governo, è arrivata a definire il superbonus, testualmente, «il più grande regalo fatto dallo Stato a truffatori». parole che, oltre a segnalare come la virtù della continenza verbale evidentemente non appartenga alla Presidente del Consiglio - ma questo l'avevamo capito - ponendo in tutta la sua evidenza il furore ideologico che ha accompagnato e accompagna la narrazione su questi temi; un furore che non ha consentito all'onorevole Meloni di capire come, con quelle parole, in un colpo solo, ha offeso imprenditori onesti, artigiani laboriosi, professionisti capaci e proprietari di immobili che sul superbonus stanno patendo difficoltà profonde e danni irreversibili. *(Applausi)*. La vera truffa, a voler evocare le improprie parole utilizzate dal Capo del Governo, sta piuttosto nella circostanza che il Governo stesso non rispetta gli accordi con i cittadini, rompendo un patto di fiducia che è alla base della credibilità delle istituzioni, della democrazia e della stessa economia. La verità è che sulla vicenda dei *bonus* edilizi si rischia, una volta di più, di incrinare il già fragile rapporto tra cittadini contribuenti e lo Stato. Se fai un patto con il Paese attraverso una legge che riconosce aiuti fiscali, non puoi in corso d'opera cambiare per ben 22 volte le norme e in ultimo cancellare quel patto, lasciando le persone fuori di casa e le imprese coperte di debiti. Allora, di fronte a tutto questo, per poter discutere con cognizione di causa del tema, servono chiarezza e verità. Punto primo: l'impatto economico complessivo del superbonus 110 per cento sull'economia nazionale, secondo vari studi, è pari a 195 miliardi di euro, dei quali con effetto diretto pari a quasi 88 miliardi, con effetti indiretti per 40 miliardi e 67,8 di indotto. Il confronto tra il 2022, anno di entrata a regime della misura, e il 2019 fa registrare un incremento di quasi il 40 per cento degli investimenti in edilizia, trainando la crescita del PIL nel 2021 e nel 2022, con l'aumento della domanda interna e con un conseguente contenimento del rapporto debito-PIL. Punto secondo: è una totale falsità che di questi bonus abbia approfittato solo una platea di redditi medio-alti per ammodernare la propria villetta. E questo non lo diciamo noi o lo dice l'opposizione, ma è l'Ufficio parlamentare di bilancio ad avere accertato che, a differenza del precedente regime di agevolazioni edilizie ed ecobonus, di cui hanno beneficiato maggiormente i contribuenti con un patrimonio immobiliare e un reddito alto, che, disponendo di liquidità e di capacità fiscale sufficiente, potevano effettivamente scomputare le detrazioni dal debito d'imposta, con il superbonus 110 lo sconto in fattura e la possibilità di cedere il credito cito ancora - consentono di superare i problemi che limitano la possibilità di fruire dell'agevolazione a quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione. È un evidente aiuto, dunque, agli incapienti fiscali. Punto

1,3 milioni di unità abitative. A fronte di una spesa agevolata di 57 miliardi, risultano entrate dirette nel bilancio dello Stato per i lavori effettuati pari a quasi 26 miliardi, ovvero il 47 per cento della spesa complessiva, derivate dai redditi Irpef per operai e professionisti, nonché dall'IVA su prodotti e forniture. A tali effetti diretti vanno poi aggiunti quelli indiretti, come ad esempio l'incremento di produzione per forniture e materiali, che consentono un aumento delle entrate per lo Stato tale da arrivare a un complessivo 75 che, per effetto del superbonus, si è registrata un'emersione di circa 150.000 lavoratori del mondo dell'edilizia che prima non erano conosciuti, con un'evidente aumento delle entrate da recupero dell'evasione. E non è l'unico recupero del sommerso: non si tiene infatti in debito conto quanto la manovra del superbonus abbia consentito di recuperare nell'ambito del patrimonio edilizio privato (un ampio numero di immobili fino a ieri del tutto invisibile). Penso a quante abitazioni, a seguito delle opere di adeguamento energetico e sismico, saranno finalmente censite, accatastate e computate nei ruoli fiscali degli enti locali, generando gettito sulla fiscalità locale, prima evaso, che si aggiunge alle percentuali già accennate. le tanto sbandierate truffe non hanno riguardato se non in percentuali minime il superbonus, ma hanno perlopiù riguardato altri *bonus*, soprattutto nella fase in cui le asseverazioni dei progettisti non erano previste quale presupposto di regolarità e utilizzabilità per le detrazioni. In particolare, ci possiamo riferire al *bonus* facciate: basti pensare che solo il 3 per cento dei crediti utilizzati per cento, mentre l'80 per cento riguarda il *bonus* facciate o l'ecobonus. I dati ci dicono dunque un'altra verità, quella autentica, su una misura che il Governo ha provato a infangare davanti all'opinione pubblica. Tutti questi dati che ci parlano di una misura positiva per il Paese sono tuttavia sufficienti a dire che andava mantenuta com'era? Per noi no. Su questo condividiamo l'osservazione che la misura avrebbe avuto e avrebbe bisogno di correttivi e migliorie; di una maggiore attenzione al controllo dei prezzi; un miglior sistema di controlli e asseverazioni; di maggiore attenzione per le fasce più deboli; di un sistema sostenibile di monetizzazione del credito per le imprese che hanno concesso lo sconto in fattura garanzie su un maggiore aumento del salto delle classi energetiche generali: tutti correttivi che avrebbero potuto essere introdotti senza sconvolgere le misure di agevolazione e l'intera filiera delle costruzioni. Il decreto-legge oggi in discussione non risolve il problema sul campo, si limita a introdurre una specie di sanatoria per coloro che non sono riusciti a completare i lavori, abdicando rispetto alle concrete soluzioni che sarebbero state necessarie; una sanatoria peraltro ulteriormente discriminatoria rispetto ai tanti che nel corso degli ultimi mesi hanno compiuto enormi sforzi tecnici ed economici per chiudere i cantieri, rispetto a chi invece non ha contratto debiti e oggi trova la via d'uscita della sanatoria. Per non parlare del contributo previsto al comma 2 dell'articolo 1, strumento sostenuto da risorse pari a 16 milioni disponibili, in grado di far fronte appena a qualche centinaia di unità immobiliari, mentre la vicenda riguarda centinaia di migliaia di immobili in tutto il Paese. Vi è poi un contributo, cioè un sostegno economico a sportello (tale per cui chi arriva prima lo prende), che rifonde pagamenti preventivamente anticipati dai proprietari, che inoltre non devono superare un ISEE di 15.000 euro per rientrare tra i beneficiari della misura. Insomma, è un vero e proprio pasticcio. Per vostra responsabilità, nelle prossime settimane saremo spettatori di gravi contenziosi e fallimenti di molte imprese. Avrete la responsabilità di spiegare loro - tanti dei quali sono vostri sostenitori ed elettori - che avete preferito la propaganda delle truffe alla politica della riconoscenza per i tanti sacrifici che hanno fatto in questi mesi con i crediti incagliati. Sarete costretti a spiegargli che cedere un credito alla metà del valore è colpa loro e delle truffe che hanno compiuto, mentre la grande colpa è di un Governo che ha incentivato e incoraggiato queste manovre speculative, ignorando le richieste di aiuto e scartando senza motivo

con un sol colpo, dichiararsi contro la transizione ecologica ed energetica, contro gli imprenditori dell'edilizia e contro le famiglie che, dopo tanti sacrifici per costruire o comprare una casa, oggi non sanno come uscirne. Che fine hanno fatto il centrodestra a difesa della famiglia, i moderati fautori dello *slogan* «la casa è sacra» e del sostegno alle imprese? Come a noi anche a voi hanno chiesto un incontro i rappresentanti della filiera delle costruzioni. Noi li abbiamo incontrati, abbiamo ascoltato l'ANCE che è l'associazione dei costruttori, Confindustria, non un'organizzazione sindacale di base. Noi li abbiamo ascoltati, voi non li avete ascoltati. Avete perso su questo e su tante altre vicende la cultura di governo e alla fine vi siete persi. I danni sui *bonus* edilizi, frutto delle vostre scelte, delle vostre omissioni, saranno gravi e ne porterete la responsabilità per anni, mentre invece dovevamo studiare insieme una misura strutturale, coinvolgendo l'Europa, magari un *next generation house*, una grande opera di infrastruttura di infrastruttura europea per le case, che sono peraltro la principale causa di incremento del caos climatico e invece non l'abbiamo fatto. Saremo qui a ricordarvelo insieme ai tanti che saranno vittime delle vostre scelte, che voi state abbandonando e al fianco dei quali noi invece vogliamo restare.

Presidente, colleghe e colleghi, con questo provvedimento, recante disposizioni in materia di agevolazioni fiscali in edilizia, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra cogliamo l'occasione per sottolineare con forza quanto sia importante introdurre e mantenere nel nostro ordinamento strumenti economici che consentano di generare per le famiglie e le imprese un concreto risparmio energetico ed economico; opportunità che purtroppo il Governo Meloni non vuole cogliere quando si tratta di contrastare efficacemente gli effetti distruttivi del cambiamento climatico. In questa direzione si era mosso il tanto criticato superbonus, misura introdotta nel 2020 con il cosiddetto decreto rilancio, oggi al centro di una irresponsabile campagna politica di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Questo Governo ha infatti deciso di perseguire la solita vecchia logica politica demolitoria, impegnandosi di fatto a smantellare per intero un efficace meccanismo di agevolazione fiscale che, al netto delle sue criticità economiche, ha comunque portato al Paese innumerevoli ricadute positive in termini ambientali, sociali e di risparmio sui costi energetici in bolletta. Ha voluto ignorare l'obiettivo principale dell'agevolazione in esame, e cioè quello di ridurre i costi ambientali ed economici connessi al consumo dell'energia, provvedendo, secondo una logica tutta italiana del fare e disfare, a distruggere di notte ciò che si era fatto di giorno, senza considerare gli effetti migliorativi che questa misura ha portato al nostro Paese: effetti concreti che, in mancanza di una politica innovativa e lungimirante di questo Governo, siamo costretti a spazzare via in una logica compulsiva, senza nemmeno avere la possibilità di valutare nel dettaglio come modificare e migliorare legislativamente in corso d'opera questo importante strumento di sgravio fiscale. Ci sono stati benefici ambientali in termini di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, risparmi economici maturati in bolletta dagli utenti finali, la creazione di nuovi di nuovi posti di lavoro. Questi sono solo alcuni degli aspetti positivi che non possono e non devono essere trascurati quando parliamo della misura del Analizzando gli impatti economici e sociali generati dal cosiddetto superbonus, è evidente come l'aumento del numero e del valore degli investimenti a questi connessi abbia contribuito a una crescita esponenziale del dato occupazionale nel breve periodo, ma abbia anche generato - come confermato anche da Bankitalia un risparmio consistente sui costi energetici per gli utenti finali; una riduzione della dipendenza energetica dall'estero - non dimentichiamolo - una riqualificazione degli edifici e, più in generale, un deciso avanzamento nel processo di transizione ecologica. Questo Governo fatica a comprendere che i benefici generati dal cosiddetto superbonus sono molteplici e interconnessi tra loro. La portata trasversale di questo incentivo ha una valenza di sistema importantissima. A livello occupazionale, per esempio, l'ANCE stima, per ogni miliardo di euro di spesa aggiuntiva nel comparto delle costruzioni, un aumento di circa 16.000 occupati. Tutto ciò senza tralasciare la riduzione dei costi della bolletta elettrica - come ho già detto - e il conseguente abbattimento delle emissioni climalteranti: obiettivo europeo che dobbiamo traguardare al più presto non solo per rispettare gli impegni presi a livello internazionale ed europeo, ma anche per salvaguardare la nostra salute, la nostra vita e il nostro pianeta. È di questi giorni la notizia che vede Milano, per la sua qualità dell'aria, come una delle città più inquinate al mondo. Da tempo, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra stiamo denunciando l'aria pessima della Pianura Padana, classificata dall'Agenzia europea dell'ambiente tra le zone più inquinate d'Europa. Al di là di qualsiasi *ranking*, ormai ce ne stiamo rendendo conto di persona di quanto pessima sia l'aria in tutto il Nord Italia. La cappa visibile delle ultime settimane sulla Pianura Padana la stiamo vedendo e respirando tutti. È lì a testimoniare quanto poco si stia facendo per contrastare l'inquinamento atmosferico, causa di patologie a polmoni, cuore e occhi; gli stessi occhi che in Italia non volete aprire per riconoscere anche le difficoltà in cui si trova il Sistema sanitario nazionale, costretto ad affrontare gli enormi costi causati dall'aumento di queste malattie. È una situazione grave e preoccupante, che ci pone seri dubbi in merito alla vivibilità di intere città della nostra penisola, ormai inghiottite dallo smog e strozzate dalle polveri sottili, principale causa delle morti premature per inquinamento atmosferico: circa 60.000 Di questo passo dove arriveremo? Sulla base dei dati registrati oggi in Pianura Padana, da sempre uno dei luoghi più inquinati del Paese, attualmente sono sconsigliate attività all'aperto, si dovrebbero tenere le finestre chiuse e bisognerebbe indossare la mascherina per gli spostamenti esterni. La mascherina, uno dei simboli dell'emergenza pandemica, potrebbe diventare un nostro quotidiano strumento di protezione, così come accade nelle megalopoli orientali. Bell'esempio che stiamo imitando. Sono questi il presente e il futuro che vogliamo avere? Lo chiedo a questo Governo che, sordo e cieco rispetto a tali problemi, continua a snobbarli e ignorare le emergenze, cavalcando in modo irresponsabile la logica politica dell'interesse e della ricompensa elettorale a breve termine. Inoltre, il Governo sta di fatto sanando situazioni di abusi edilizi, continuando a ragionare e ad agire secondo una logica di un mondo che non esiste più, mostrandosi restio nell'attuare quelle politiche di adattamento e di mitigazione del cambiamento climatico, che riducono efficacemente i consumi energetici e contribuiscono ad abbattere gli impatti gli impatti ambientali a partire dal primo mattone che si posa in una costruzione. Com'è possibile non aver capito che oggi non ci possiamo più permettere di costruire senza prevedere il rispetto di criteri minimi ambientali obbligatori, che possano salvaguardare e garantire un minore impatto ambientale di tutti gli edifici? Ad oggi dobbiamo prendere atto che il problema dell'abusivismo edilizio ha portato, in molti casi, a veri e propri disastri. Interi ecosistemi ambientali e ricchi di biodiversità sono stati devastati al cospetto di scheletri di cemento fatiscenti, mostri edilizi orripilanti. È inaccettabile andare sempre alla ricerca di qualche capro espiatorio e non cogliere l'opportunità di una discussione costruttiva. All'interno della stessa maggioranza, nel surreale dibattito svoltosi alla Camera su questo provvedimento, c'è chi ha compreso le problematiche in essere e la necessità di un cambio di passo nel comparto dell'edilizia e chi, invece, non ha manifestato alcun interesse a tutelare i diritti di persone, imprese e ambiente. Tant'è che anche qui sono stati presentati alcuni emendamenti contraddittori da parte delle forze politiche della maggioranza. Garantire il rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, richiede un comportamento maggiormente responsabile, più coraggioso e innovativo, che purtroppo manca al Governo Meloni e manca a questo provvedimento.

il presidente Meloni tuonava che eravate pronti, prontissimi a difendere i diritti delle imprese edili, dei lavoratori dell'edilizia; pronti ad aiutare le imprese con i crediti incagliati. La Lega e Salvini dichiaravano che il superbonus aveva fatto crescere enormemente l'edilizia. Forza Italia voleva estendere il superbonus in tutti i settori. Quindi, la vera truffa non è il superbonus. La vera truffa è quello che avete promesso in campagna elettorale nell'autunno del 2022, perché questa è l'ennesima promessa che avete fatto agli italiani e vi siete rimangiati. Voi avete parlato chiaro alle imprese edili. Avete fatto delle promesse ben chiare e oggi attaccate le stesse imprese edili, che si vedono appunto ingannate dalle vostre promesse. Riconoscete almeno il fatto e cercate di rivedere quello che avete detto in campagna elettorale, dove avete promesso di tutto e di più. Quella è la grande truffa che avete fatto a questo Stato e ai cittadini italiani. Il superbonus è una misura che ha avuto una rilevanza enorme nel nostro Paese; una misura pensata e attuata da luglio 2020, in piena pandemia, quando l'economia italiana era praticamente ferma. I continui *lockdown* avevano creato uno uno stop di tutte le attività imprenditoriali e quindi serviva qualcosa, un po' come quando un paziente ha un infarto. Il

a un settore trainante come l'edilizia, un settore che fa lavorare tantissime persone e che include almeno venti indotti, dalla ceramica all'idraulica, a tantissime altre attività che vengono svolte nel nostro Paese. Il superbonus ha avuto il Governo Conte ha pensato questa misura proprio per diciotto mesi, dal luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Considerate che il Governo Conte è caduto il 26 gennaio 2021;

il costo del superbonus era di 16 miliardi. Quindi, colleghi, non potete imputare al Governo Conte i costi di questa manovra. Dal momento in cui il Governo Conte è caduto ad oggi, il superbonus ha subito ben 33 modifiche. *(Applausi)*. Quindi, è un'altra legge: è stata trasformata dal Governo Draghi, che di edilizia non ne sapeva nulla, ma gli interessi delle banche li sapeva fare, perché, incagliando i crediti, le banche non scontavano più al 105, ma scontavano all'85. *(Applausi)*. Quindi, il Governo Draghi i profitti dell'edilizia alle banche (extra profitti che voi non avete tassato). Il Governo Draghi edilizia non ne sapeva nulla e, infatti, ha confuso il superbonus con il bonus facciate, facendo una figura

cento di quanto speso nel superbonus ritorna il primo anno (questa è la stima peggiore). Quindi, se è vero che è costato nella sua vita 100 miliardi, la stima peggiore ci dice che almeno 43 miliardi sono rientrati nel 2022, quando governava Draghi. Dove sono finiti i 43 miliardi? *(Applausi)*. Si sono spesi quasi 100 miliardi per combattere la crisi energetica causata dalle guerre. I soldi del superbonus li avete spesi. Questi sono i dati del bilancio. Si è pagata la crisi energetica, tagliando i costi delle bollette, e questa misura è costata oltre 50 miliardi; avete preso i soldi del superbonus per pagare la crisi energetica causata dalle guerre. dalle guerre. Gli incassi del superbonus, invece di destinarli alle imprese che hanno operato onestamente, li avete spesi per altri motivi. Questo è ciò che è successo. Quindi c'è un superbonus del Governo Conte che è costato 16 miliardi, un superbonus del Governo Draghi che è costato circa 40 miliardi, i cui incassi sono stati poi utilizzati per la crisi energetica, e poi c'è un superbonus - voi governate da oltre un anno e mezzo - gestito malissimo da questo Governo, perché non è stato capace di creare una misura di lungo raggio. È vero, infatti, che il superbonus al 110 per cento serviva in quella fase di pandemia, ma è pur vero che serviva una misura di medio-lungo periodo. Dopo l'elettroshock causato dalle pandemia e risolto dal superbonus, serviva una politica di medio-lungo periodo per consentire di raggiungere quegli obiettivi che l'Unione europea ci ha chiesto, ma voi non siete stati capaci di farlo. Era fondamentale, dai primi mesi di questo Governo, lasciare il 100 per cento per chi non ha nulla, per chi non è in grado di restaurare la propria casa, perché non hai i soldi per farlo, e prevedere per chi ha la possibilità di farlo grazie a dei redditi più consistenti. Dovevate fare questo un anno e mezzo fa, perché non l'avete fatto? *(Applausi)*. Ora vi lamentate che il superbonus incide sul bilancio: perché quando siete arrivati non avete fatto una misura di *décalage*? *décalage*? Noi abbiamo finito di governare il 26 gennaio 2021, ultimo giorno del Governo Conte. Sono passati oltre tre anni

e avete ingannato le imprese edilizie, a cui avevate promesso di mantenere il superbonus. Pertanto il vero fallimento è vostro, della vostra politica che non è capace di fare nulla. Siete capaci solo di criticare e di trovare scuse per dire che non state riuscendo a mantenere le promesse che avete fatto in campagna elettorale. Adesso è caduta l'ultima scusa, non ne avete più; da un anno e mezzo fa fino ad oggi avete detto che non avete varato

quello che è stato fatto dai Governi precedenti, ma qual è la vostra visione? Quali sono le vostre misure? Cosa volete fare per far crescere l'economia di questo Paese? Basta con questi piagnistei, iniziate a dirci voi cosa siete in grado di fare. Noi lo abbiamo detto. In fase di pandemia abbiamo fatto crescere l'economia e abbiamo portato oltre 200 miliardi del PNRR, di cui vi state vantando.

io su questo sono d'accordo, perché gli obiettivi che l'Unione europea ci dà sono ambiziosi: abbiamo bisogno di risanare le nostre case. Avete visto l'inquinamento nella Pianura padana.

tecnologie altamente efficienti che portano energia pulita, le stesse che incentivava il superbonus, che è stata una misura importantissima per il nostro Paese, ma che è stata rovinata da 33 modifiche e dal fatto che non siete stati capaci

che rappresentano 60 milioni di italiani e su tanti provvedimenti, in un Paese che ha conosciuto il tempo del Rinascimento e del Risorgimento, bisogna essere sempre molto responsabili. Che cosa è il superbonus? Ci ascoltano anche delle

quale la politica, votando, assume la responsabilità dei provvedimenti. Ogni provvedimento ha una sua epoca storica. Per quanto riguarda le spese fiscali, i *bonus* e quant'altro, c'è una visione sostanzialmente differente. Quando sono arrivato in Parlamento e ho iniziato a lavorare in Commissione finanze, immaginavo che avessimo circa 300-350 spese fiscali, cioè una moneta parallela. Dico agli moneta parallela. Dico agli ultimi che sono intervenuti, con grande rispetto, perché ciascuno di noi rappresenta una umanità che è professionale, familiare ed anche politica e ideale: ci piacerà ricordarvi sempre su quel balcone, con la vostra convinzione di aver abolito la povertà *(Applausi)*; quella è l'immagine

quelli con cui ho vissuto una vita istituzionale a livello regionale e anche oggi in Parlamento, e penso quanto sia importante che ci sia un contrappeso a delle valutazioni estremamente tecniche su cui un Governo politico si gioca la faccia. Un Presidente del Consiglio e i Ministri fanno delle scelte

il lascito ricevuto. Voglio fare un passaggio sui toni del nostro collega del PD e sul richiamo alla responsabilità. I fantocci per strada, la divisione ideologica, hanno portato in tanti anni a un'Italia che non ci piaceva. Mi riferisco anche al racconto di alcuni giornalisti. Ho visto tante volte facce di politici grazie a Dio, ci sono stati quelli di centro, di destra e di sinistra - e i faccioni sui giornali, nella stagione che ha portato quelli di uno vale uno - che tutti insieme non valevano nulla - ad abolire quasi il Parlamento. Tutti sapete quanta difficoltà c'era a lavorare in Commissione, perché nel loro racconto c'era un'Italia che non funzionava

trasferirvi quanto è complessa la nostra funzione e quanto le due visioni siano oggettivamente diverse. Noi rivendichiamo la nostra. Chi è seduto qui,

sappiate bene che l'avverbio migliore che utilizzerà non sarà gratuitamente, ma sarà responsabilmente. *(Applausi)*. Questa è la differenza sostanziale quando si guarda al proprio popolo, alla Nazione e si cerca di mettere in campo gli strumenti

Voi siete il concepimento giusto e legittimo, nessuno lo mette in discussione perché amiamo la democrazia, così come amiamo quell'importante consenso che ha portato questa maggioranza con la sua sensibilità oggi a governare il nostro Paese; siete il prodotto di una Nazione e quindi di tanti Governi tecnici (dai fondi internazionali, da quell'Europa, che ovviamente noi agognavamo come Europa dei popoli e che non ci piace perché oggi vogliamo cambiare). Ecco, questa è la sintesi del dibattito oggi in Parlamento. Un provvedimento che non avete nemmeno l'intelligenza - ribadisco - non il coraggio, di stabilire che non ha funzionato,

e altro) circa 300 ville e cinque castelli. Se non si ha il senso della misura sul risultato di questo provvedimento, fatto con tutta la buona fede possibile, se non valeva nulla Conte, magari non valevano molto i tecnici che hanno suggerito questo provvedimento, che ha necessità del trentesimo intervento

crediamo ci sarà un tempo che magari gli italiani vogliono provare un'altra visione e un altro Governo - a costruire riforme di medio lungo periodo. al nostro esame non si legge soltanto nell'intervento di andare a mitigare un danno; doveva valere 20 miliardi all'anno ed è arrivato a 60-70 miliardi, con un buco che ha fatto saltare le politiche di bilancio per questo Stato per tanti anni a venire. Bene quindi che ci sia adesso il PNRR e che ci siano gli altri investimenti. Si sta realizzando in questo momento - e su questo ci piacerebbe avere un confronto - in contemporanea la riforma orizzontale e verticale dello Stato, le autonomie, il premierato, l'autonomia differenziata, la riforma Proviamo ad elevare il dibattito, anche rispetto all'utilizzo delle parole. Nulla accade per caso: le lettere, i proiettili, i fantocci che vengono accesi per strada,

Presidente, per il suo tramite mi scuso per il mio fuori onda, ma era per stabilire quanto, come e perché responsabilmente non riescono a dissociarsi dalla vicenda che abbiamo vissuto nel fine settimana, quella di chi di incontinenza verbale, quasi al limite della demenza, sporca le istituzioni e noi in queste istituzioni, più che gratuitamente, vogliamo continuare a starci responsabilmente.

degli interventi più variegati, l'uno in contrasto con l'altro, la difficoltà reale che si è incontrata affrontando questo argomento è data dalla natura di quello stesso provvedimento, che è vero che nella fase iniziale poteva avere un suo perché, dato dal fatto che c'era la necessità di rilanciare un percorso, ma è un provvedimento nato male,

ben intendere quello che si voleva ottenere facendo un provvedimento di questo genere, sapendo benissimo quale strascico avrebbe portato dietro. C'è stata una difficoltà reale che stiamo tentando di gestire nel miglior modo possibile, perché abbiamo un'idea di sviluppo del nostro Paese che va in in una direzione completamente diversa rispetto a quello che è stato fatto fino ad ora. Rispetto a questo mi sembra evidente che ci siano una direzione e un indirizzo completamente diversi. C'è necessità di farlo con il tempo, perché non abbiamo la bacchetta magica, evidentemente, in una fase come questa, ma è logico che l'indirizzo che è stato intrapreso e tutti i parametri economici ci lasciano intendere che siamo sulla strada giusta. La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e continueremo a portarla avanti per l'intera legislatura e per la prossima.

del superbonus avevano con sé anche l'installazione dei pannelli fotovoltaici. Sia il risparmio energetico agevolato dalla copertura, dalla coibentazione degli edifici, che ha procurato un risparmio nella richiesta di energia, sia la produzione di energia attraverso i pannelli fotovoltaici hanno portato chiaramente dei vantaggi, che però non vengono contabilizzati. Quindi, questo ordine del giorno chiede al Governo di attivarsi al fine di individuare e di adottare misure a rendere di pratica e concreta attuazione il calcolo dei risparmi generati dagli impianti fotovoltaici e dai sistemi di accumulo installati grazie alla misura del superbonus nella fattura energetica nazionale del 2022, con riferimento alle minori importazioni di petrolio e di gas e alla riduzione delle emissioni di CO2 e ad includere tali risultati nei rapporti di ENEA e degli altri enti nei prossimi anni. Stiamo parlando di circa tre miliardi. Ora, è chiaro che se vogliamo instaurare un metodo, se vogliamo osservare la situazione, dobbiamo raccogliere i dati e contabilizzarli, altrimenti sarà difficile pianificare la direzione in cui l'Italia vuole andare ai fini del risparmio energetico e della produzione autonoma di energie rinnovabili. Mi fa specie che questo Governo non abbia accolto questo ordine del giorno, perché si tratta semplicemente di trasparenza, di rendicontazione utile alla pianificazione futura. Ma forse questo Governo non sa bene da che parte pianificare.

Signor Presidente, questo ordine del giorno fa seguito ad un impegno che il Governo aveva assunto, in fase consultiva in Commissione finanze alla Camera, circa la volontà di rimediare con una disciplina organica all'evidente disparità creatasi tra due tipologie di cittadini e di contribuenti: cioè chi, in una fase in cui non era in grado di prevedere questo intervento normativo, aveva optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Come sapete, il decreto che stiamo votando segna una netta demarcazione tra queste due tipologie di cittadini, che avevano un affidamento riguardo al legislatore e agli impegni del Governo. Ci era sembrato di cogliere un'apertura su questo fronte e quindi riproponiamo questo ordine del giorno, chiedendo un impegno per lo meno a limitare questa disparità, così come ci era sembrato di cogliere nel lavoro di Commissione.

Presidente, su questo ordine del giorno, che fa riferimento ad un caso specifico avvenuto a Roma, a Colli Aniene, dove un'intera palazzina è stata distrutta da un evento imprevedibile avverso, come un incendio, mi sembrava di aver colto una disponibilità in Commissione da parte del Governo con una riformulazione, quindi con un invito più tenue, che noi saremmo disposti ad accogliere, se il Governo confermasse in questa sede la stessa disponibilità mostrata in Commissione.

Presidente, colleghi, oggi all'esame dell'Assemblea c'è un provvedimento che riguarda i cosiddetti *bonus* edilizi. Questa maggioranza non si è mai posta pregiudizialmente contraria a sostenere, anche attraverso lo strumento degli incentivi fiscali, il settore dell'edilizia. Anzi, per noi è stato sempre essenziale sostenere un comparto che è traino della nostra economia nazionale. È evidente però che si rendeva necessario porre rimedio agli errori del passato in merito soprattutto ad una sottovalutazione delle coperture economiche di queste misure. vero infatti, come è vero, che con un costo di 140 miliardi abbiamo riqualificato il 4 per cento degli edifici italiani, questo significa che, per riqualificarli tutti, avremmo dovuto spendere 2.500 miliardi di euro, una cifra chiaramente enorme e sproporzionata. Il superbonus è stato costruito male e, così come è stato concepito, è stato uno strumento insostenibile Forse si sarebbe dovuto riflettere fin dall'inizio su interventi più razionali e selettivi. E invece qual è il messaggio che è passato nella testa dei nostri cittadini? Si poteva ristrutturare gratuitamente la casa, senza magari dedicarsi troppo ai preventivi. È chiaro che è passato un messaggio sbagliato che, anziché sostenere il comparto dell'edilizia, portando ad una spesa fuori controllo, ha finito per danneggiare questo comparto e tutto il mondo dell'artigianato e dell'impresa che a noi stanno particolarmente a cuore. Questo spreco di denaro pubblico ha fatto delle vittime; *in primis* i proprietari delle case, i nostri cittadini che sono rimasti nel limbo dell'incertezza normativa per tanto, troppo tempo, così come i professionisti, le imprese e il sistema bancario che si è ritrovato ad avere in cassa crediti cosiddetti fasulli. Va detta però una cosa: se una legge è sbagliata, è giusto non far ricadere sulle spalle di un contribuente le sue conseguenze. Ecco perché Ecco perché nell'ultima legge di bilancio abbiamo stanziato, ad esempio, 20 miliardi per consentire il completamento delle opere a chi è arrivato a un certo punto nell'utilizzo di questo superbonus. Correggere gli errori del passato: questa è la *ratio* del provvedimento. La riprova sta in un numero: su 140 miliardi di superbonus 12 miliardi sono di frodi certificate. È il segnale che c'era qualcosa che non andava. Ecco perché era necessario modificare in corsa le regole. In un provvedimento precedente, ad esempio, abbiamo messo in sicurezza il terzo settore nel sistema sociosanitario, perché abbiamo previsto che il 110 per cento fosse coperto fino al 2025.

Anziché fare la politica degli *slogan* e del *marketing*, abbiamo preferito la politica della concretezza e delle soluzioni fattibili. Noi preferiamo la concretezza, dare risposte concrete ai cittadini, anziché dare illusioni e gettare fumo negli occhi, magari solo per ottenere un *like* sui *social* o qualche consenso in più. *(Applausi)*. Questo è lo spirito del decreto-legge che andiamo a votare oggi. Ecco perché annuncio il voto favorevole al provvedimento del Gruppo UDC-Noi Moderati-Coraggio Italia-MAIE.

dopo circa un anno e mezzo siamo finalmente arrivati, anzi siete arrivati, alla resa dei conti sul superbonus. Per oltre un anno questo Governo ha adottato una tattica attendista, dilatoria, affrontando il tema del superbonus in maniera sempre laterale, cercando di scansarlo e di rinviarlo. In legge di bilancio a dicembre, circa un mese e mezzo fa, siete quasi arrivati a litigare all'interno della maggioranza, perché Forza Italia Italia reclamava la difesa dei patti e degli accordi e il resto del Governo, invece, continuava a negare e rinviare. Questo rinvio alla fine è giunto al termine. Questa partita sul superbonus va definita e conclusa, come vediamo in questo testo che ci arriva preconfezionato, sul quale il Governo non ha voluto che venisse apportata alcuna modifica, che ha blindato con un secco no a qualsiasi richiesta, anche la più più ragionevole, anche quella che non avrebbe comportato aumento di spesa. E questo la dice lunga sull'approccio che questo Governo ha sulle misure rivolte alle famiglie; quelle famiglie che dite di voler aiutare e sostenete di aiutare e che invece gravate con imposizioni continue e con l'aumento delle imposte indirette, che sono la peggiore imposizione possibile in economia, perché sono quelle che colpiscono tutti, indipendentemente dalla fascia di reddito. E lo fate aumentando l'IVA sui prodotti dell'igiene femminile, aumentando l'IVA sul latte in polvere, aumentando l'IVA sui seggiolini per i bambini e rendendo sempre più difficile l'Opzione donna, riconoscendo un *bonus* mamme soltanto alle donne che hanno più di due figli, perché sotto due figli non si è abbastanza mamme per questo Governo o addirittura non si è abbastanza donne e, quindi, non si dà proprio nulla. *(Applausi)*. Ecco che col superbonus la fate completa e scaricate sul peso delle famiglie l'ultimo

Ed è nata anche con l'obiettivo di coniugare questo intervento con un altro progetto, una finalità sicuramente elevata, che è quella di efficientare il patrimonio immobiliare italiano e di dare delle risorse per mettere finalmente patrimonio immobiliare in condizioni di essere *green*, di fare una transizione energetica e di abbattere le barriere economiche, cioè fare un investimento che non fosse una speculazione immobiliare, perché non lo era. Non era questo nelle visioni e nelle iniziative, quando venne concepito

Con esso si spiega per quale ragione il cittadino, quando accetta una norma dello Stato, per esempio quando stipula un accordo, sottoscrive un impegno o - come in questo caso - presenta domanda per ottenere un superbonus, ha diritto

e ancora una volta a discapito delle fasce di reddito più in difficoltà *(Applausi)*, delle famiglie e anche delle imprese. Il grande problema del superbonus nasce quando il ministro Giorgetti, arrivato in Aula all'inizio di questa legislatura, interrogato proprio sulla vicenda del superbonus, che aveva determinato una situazione di stallo nell'edilizia, uno dei settori trainanti dell'economia italiana,

che avevano dato in appalto a un'impresa i lavori con il superbonus avessero diritto a vedere riconosciuto questo credito ceduto all'impresa; era una facoltà. era una facoltà. E nel momento in cui si dice che è una facoltà, lo Stato abdica al suo ruolo e non è più garante di un patto tra lo Stato, le famiglie e le imprese, riconducendolo a una dimensione negoziale e privata, a un accordo tra le banche e tra le imprese, che può essere sottoscritto, ma anche rifiutato.

Cosa sono i crediti incagliati? Sono soldi immaginari, sostanzialmente, che teoricamente ci sono, perché le famiglie hanno affidato l'esecuzione dei lavori alle imprese, che si sono impegnate ad eseguirli per un valore che è stato approvato. E questo credito è stato iscritto alle banche: è stato chiesto di trasformarlo in un credito effettivo e le banche si sono rifiutate; non è che il credito non esista più, ma è incagliato. È un'espressione paradossale, come quelle dei film: i soldi dove sono? Sono incagliati. Ma io li ho? No. Li posso spendere? No. Li posso disincagliare? No: paradossalmente, neanche questo si è potuto fare. Perché? I direttori di banca rispondevano: perché aspettiamo una risposta dal Governo, se li possiamo o no restituire, almeno virtualmente, o li dobbiamo tenere incamerati. Oggi il Governo risponde, finalmente: almeno,

modo, la misura del superbonus 110 per cento viene riconosciuta a chi ha raggiunto una quota di lavori non inferiore al 60 per cento entro il 31 dicembre 2023. In questo caso il decreto riconosce un contributo soltanto ai cittadini che abbiano un reddito non superiore a 15.000 euro in relazione alle spese sostenute dal primo gennaio fino al 31 ottobre 2024. Cosa vuol dire in parole povere questa misura? parole povere questa misura? Significa che io prendo i crediti che ho maturato nell'esercizio precedente, li riconosco nell'esercizio attuale, ma dico anche che intanto ne puoi usufruire soltanto se sei in una condizione di fascia di reddito bassa, e poi aggiungo che, siccome verosimilmente non ne potrai neanche usufruire, perché non ce la farai a stare in questi parametri, questo vantaggio, che voleva essere una misura per rilanciare l'economia e per aiutare le famiglie, finirà per essere inesigibile. Siamo cioè passati dai crediti incagliati ai crediti inesigibili, di cui le famiglie non potranno più beneficiare, non se ne faranno nulla. In conclusione, Presidente, che dire del fatto che il contributo viene erogato soltanto per la sanatoria e soltanto fino alla disponibilità dei fondi, cioè soltanto fino alla capienza di 16,4 miliardi. È una misura veramente minima, iniqua, davvero evidentemente insufficiente per poter completare la vicenda del superbonus e per poterla concludere in modo tale da poter dire che si soddisfa l'esigenza, la *ratio* per la quale era nato il superbonus. Invece, quando si mettono misure limitate, cosiddette fino a capienza di disponibilità delle risorse, è come se si dicesse che chi prima arriva meglio alloggia e tutti gli altri non ci interessa che fine fanno. Per questa ragione, signora Presidente, noi chiaramente su questo provvedimento non possiamo esprimere un voto favorevole e ci asteniamo.

ci sono i destini di migliaia di persone coinvolte, delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini, che hanno iniziato i lavori e hanno preso degli impegni, che in totale buona fede hanno fatto affidamento sulle misure stabilite e ora vivono il terrore di andare sul lastrico per le vostre scelte. Quindi, si è deciso di porre fine alla misura. Dovere del legislatore è trovare, però, il modo di uscire dalla agevolazione in modo ordinato, senza arrecare danni alle persone perbene. Anche sui dati non c'è stata chiarezza: troppa era l'urgenza di fare apparire questa misura uno spreco, una truffa, uno sbaglio del Governo precedente. Da maggio 2020 a febbraio 2023 risulta che si sia usufruito di 75 miliardi di detrazioni per il superbonus che il PIL sia aumentato di circa 40 miliardi l'anno. L'effetto della nuova norma è stato pertanto di circa 40 miliardi l'anno di lavori di lavori aggiuntivi, che hanno raddoppiato i volumi economici di crescita del settore costruzioni. Questo è un dato generalizzato che non dico io, ma che riporta l'associazione degli imprenditori, cioè l'ANCE. La norma ha contribuito all'incremento del PIL nazionale per una quota del 2 per cento e, a seconda dei dati di contabilità nazionale, il contributo degli investimenti in costruzioni residenziali alla crescita del PIL nel biennio scorso è stato di due punti percentuali. sarebbe riferito allo *stock* positivo generato dall'incentivo fiscale. Oltre questo c'è l'indotto, perché poi non si tratta solo di un fatto diretto; sappiamo tutti quanto sia Al di là dei dati, quindi, credo che sarebbe stato doveroso fare un passo indietro dallo scontro ideologico e un passo in avanti per cercare di entrare nel concreto di una discussione che avrà conseguenze economiche, macroeconomiche, sociali e occupazionali, e che già adesso riguarda molte persone in grande difficoltà, in condizioni di fragilità che vivono le scelte che stiamo portando avanti, che state portando avanti, con una profondissima preoccupazione. Credo che capiti anche a voi di veder arrivare, nella propria posta, centinaia, se non migliaia, sollecitazioni ad affrontare questo tema, ormai da un anno e mezzo.

che consentisse di agire in modo deciso sull'efficientamento energetico degli edifici. Sarebbe stato importante immaginare di prorogare la misura per consentire la conclusione dei lavori nei condomini IACP, così da completare il risanamento di un patrimonio edilizio che ben difficilmente potrebbe essere riqualificato in assenza di incentivi. In particolare le residenze popolari le residenze popolari sono edifici che presentano il maggior bisogno di interventi per il risparmio energetico. E gli incentivi sono un sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Sarebbe stato doveroso alzare da 15.000 a 25.000 euro il reddito di riferimento per l'erogazione del contributo previsto, per venire incontro a quei cittadini che si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà. Sarebbe, infine, stato importante - e ci era sembrato vi fosse una visione sostanzialmente condivisa - intervenire sul territorio dei Campi Flegrei, prevedendo uno speciale prevedendo uno speciale sisma bonus per i territori soggetti a fenomeni di bradisismo, che sarebbero quelli dei Campi Flegrei e anche altri. Si sarebbe dovuto e potuto intervenire per mettere in sicurezza il nostro Paese. Noi continuiamo a dirlo Noi continuiamo a dirlo in modo inascoltato e penso che il dissesto idrogeologico del patrimonio del nostro Paese, sottoposto a *stress* a causa non solo della storica presenza di eventi sismici e di vulcani, ma anche dei cambiamenti climatici in atto, sia sotto gli occhi di tutti. Quale occasione migliore per modificare in meglio, dunque, per intervenire sulla normativa, indirizzare gli interventi davvero necessari per la messa in sicurezza degli edifici,

questi mesi - è il sesto intervento al riguardo - avete continuato a mettere delle toppe, che però non hanno risolto il problema dei crediti incagliati e hanno messo in difficoltà molte imprese. Vi sono molti cantieri che non finiranno mai. Infine, avete fatto una misura che è esattamente diversa e che mette in discussione la stessa impostazione. In sostanza, avete condonato la possibilità di chiudere senza dimostrare che c'è stato l'intervento, dal punto di vista sia della ristrutturazione che del contenimento energetico. Bel risultato! In sostanza, quelli che si sono comportati in modo corretto vengono penalizzati, mentre quelli che si comporteranno in modo scorretto verranno premiati.

la misura del superbonus 110 partorita dalla creatività ideologica del MoVimento 5 Stelle, è nata male, che è risultata impossibile da salvare. misura che si basa su un pensiero scriteriato: lo Stato dà ai cittadini il 10 per cento in più di quello che spendono. Mai visto sul pianeta. misura ha introdotto la cessione dei crediti, che ha causato la più grande stortura finanziaria mai vista in materia di detrazioni fiscali, causando danni e fallimenti di imprese. Doveva essere un aiuto alle imprese del settore dell'edilizia, in crisi per la pandemia, ed efficientare il patrimonio edilizio italiano. Effettivamente all'inizio ha dato respiro e slancio al settore dell'edilizia, che però ha poi dovuto soffrire e pagare le storture della stessa misura. Nel settore si è creata anche una grande confusione, perché si sono rese necessarie decine di correzioni al disastroso impianto iniziale prodotto dal Governo Conte 2.

Inoltre gli immobili efficientati sono una percentuale risibile del patrimonio immobiliare italiano: meno del 4 per cento degli edifici residenziali ha usufruito del 110, rendendo flebile l'effetto di efficientamento energetico degli edifici e minimo l'impatto sulla riduzione dell'inquinamento. Se avessimo aiutato diversamente l'edilizia ed investito 100 miliardi in impianti di produzione di energia rinnovabile, avremmo sicuramente ridotto l'emissione dei *greenhouse* *gas* in maniera più sensibile. Perché lo Stato ha quindi speso più del previsto e ha efficientato di meno? La non stabilità di medio periodo del bonus ha creato una fretta nel sistema dei condomini, dei professionisti e delle imprese, che ha fatto aumentare la domanda; ciò ha avuto come effetto l'irreperibilità di ponteggi e materiali, con conseguente aumento spropositato dei prezzi; la nascita di migliaia di imprese senza esperienza; l'abbassamento della qualità dei lavori; le truffe; l'assenza di controllo e selezione da parte dei condomini. Sappiamo che i condomini andavano in assemblea e dicevano: «Amministratore, l'importante è che mi garantisca che non spendo un euro, poi fate quello che volete». Questo è quello che capitava nei condomini. L'aumento dei prezzi, erroneamente non previsto in fase di strutturazione della legge, insieme all'iniziale facilità con cui si otteneva la cessione del credito hanno reso ridicola la previsione iniziale di 40 miliardi di euro, portando il totale degli investimenti ammessi a detrazione al 31 dicembre 2023 a 107 miliardi, di cui 15 bloccati per verifiche su sospette truffe. Tutto questo ha creato un serio problema ai conti pubblici. Forza Italia è più volte intervenuta per aiutare le famiglie, le imprese, i professionisti e gli artigiani, onesti e in buona fede, che hanno avuto la sola colpa di credere a una legge dello Stato. Vi ricordo gli interventi che abbiamo promosso fin dall'inizio di questa legislatura, ad esempio la proroga dei termini di presentazione della CILAS. Oggi siamo stati nuovamente protagonisti nell'aiutare chi si è trovato in mezzo al guado, mediando e trovando un equilibrio tra aiuti e disponibilità finanziarie, che ricordo essere ridotte sia dal buco del superbonus che dall'enorme sforzo che questo Governo e il Governo precedente hanno fatto per aiutare imprese e famiglie a compensare l'aumento del costo dell'energia per colpa della guerra in Ucraina. E questo è un merito. Ho sentito qualcuno quasi accusarci del fatto che abbiamo dato questi aiuti. È un merito: abbiamo salvato l'economia e le famiglie di questo Paese, dando più di 100 miliardi, in un anno e mezzo, a famiglie e imprese. in esame evitiamo che il mancato completamento degli interventi del superbonus provochi la revoca dei benefici già erogati. Ho sentito anche in quest'Aula dire

sarebbe più potuto più accedere alla cessione del credito. Il problema delle truffe senza controlli avveniva all'inizio del superbonus, tre anni fa, non avveniva più in questo momento. Abbiamo aiutato le famiglie meno abbienti, riconoscendo a chi ha un reddito sotto i 15.000 euro un contributo per compensare la riduzione del *bonus* dal 110 per cento dell'altro anno al 70 per cento condomini la possibilità di concludere i lavori, perché nei condomini ci sono diverse possibilità economiche familiari: chi, messo a conoscenza del problema, potrà

che ha funzionato dal 1999, consentendoci di ristrutturare il patrimonio edilizio italiano sostenendo l'economia del settore edile in modo stabile. Basta cessione di crediti: il condomino paga l'intera somma e poi detrae una percentuale delle tasse. Questo incentiva lo stesso condomino o il condominio a scegliere con cura i professionisti, a vagliare le imprese. Torniamo a premiare chi possiede qualità ed esperienza nel settore dell'edilizia e a garantire ai cittadini di non trovarsi, come oggi, davanti all'incubo di dover pagare migliaia di euro per completare i lavori quando pensavano di averli gratis. Dovremo sviluppare un sistema di *bonus* stabile nel tempo, che garantisca alle imprese e ai cittadini una pianificazione degli interventi, soprattutto quelli di efficientamento energetico, pianificazione temporale eviterà l'aumento dei prezzi. Dovremo aiutare le famiglie meno abbienti o che non hanno capacità fiscale per le detrazioni a stare al passo con le altre, evitando di creare condomini di serie A e condomini di serie B. Dovremo lavorare perché l'efficientamento energetico sia percepito come un'opportunità piuttosto che un obbligo, come vorrebbe una parte dell'Europa. Dovremo integrare, con un grande piano di rigenerazione urbana, gli investimenti privati con quelli pubblici, per rendere le città più a misura d'uomo ed ecosostenibili. In sintesi, per sapere quale strada dobbiamo percorrere, sapendo che quella ideologica tracciata dai 5 Stelle ha portato al disastro del superbonus al 110 per cento, basta girarsi e guardare dall'altra parte. Ecco, quello è il futuro.

Governo, onorevoli colleghi, il tema in discussione è stato ampiamente dibattuto e profondamente già sviscerato in tutti i suoi aspetti, sia sul piano politico che sul piano economico. economico. Oggi abbiamo ascoltato una serie di dichiarazioni che sono prive di fondamento e io cercherò, nel breve tempo a disposizione, di fornire delle risposte su alcuni aspetti. Innanzitutto faccio una premessa e mi chiedo con quali strumenti si pensa di affrontare la transizione ecologica. Oggi l'Europa e il nostro Paese sono chiamati ad affrontare una vera e propria rivoluzione, che non è solo di carattere industriale, ma è una rivoluzione di sistema che coinvolgerà tutti: le imprese, ma anche i cittadini e quindi le famiglie. Oggi noi abbiamo la necessità di introdurre, per realizzare la transizione ecologica, dei nuovi strumenti di finanziamento che l'Europa e i singoli Stati devono fornire. Di contro, però, oggi abbiamo il Governo e la presidente Meloni che ripetono continuamente che la transizione ecologica non deve essere ideologica, ovvero

dove prendiamo i tanti soldi e le tante risorse necessarie per realizzarla e per non farla diventare ideologica, dato che il Governo ha innanzitutto accettato passivamente la iattura del Patto di stabilità imposto da Francia e Germania e dopo di che sta continuando a perseverare in una politica di austerità che impedisce, a questo punto, che la transizione ecologica non sia ideologica? I *bonus* edilizi, in particolare il superbonus, nascono proprio per realizzare la transizione ecologica e noi siamo stati pionieri, per realizzare e raggiungere gli obiettivi del PNRR, del *green new deal*, anche per affrontare le tematiche prossime che arriveranno dalla direttiva europea sulle case *green*. *green*. L'Italia è stata il primo Paese ad introdurre non solo una misura come il superbonus 110 per cento, ma soprattutto a introdurre uno strumento tecnico rivoluzionario, che è la cessione dei crediti d'imposta. *(Applausi)*. È questo lo strumento che va difeso per realizzare la transizione ecologica. Il collega che mi ha preceduto diceva: no ai *bonus*, dobbiamo ritornare alle detrazioni fiscali. Il collega forse non sa che la cubatura di quelle agevolazioni è stata minima e non è stata per nulla utilizzata; è stata utilizzata solo per chi aveva capacità fiscale, lasciando fuori tutta una serie di cittadini che vivono peraltro in quelle abitazioni non di lusso e che non si potevano permettere l'accesso al credito, di anticipare le spese, di realizzare quella transizione ecologica. Adesso mi limiterò semplicemente ad accennare ad alcuni benefici dello strumento della cessione dei crediti fiscali. Innanzitutto evidenzio gli effetti economici moltiplicatori differenti rispetto alla detrazione: detrazione: ciò permette a tutti i cittadini e a chi non ha la capienza fiscale di utilizzare l'agevolazione per la transizione ecologica, ed evita soprattutto ai cittadini di indebitarsi, con conseguente pagamento di interessi. È chiaro che oggi la maggioranza e il Governo fanno un ennesimo favore al sistema bancario, che lucrerà sull'indebitamento e sugli interessi, che oggi peraltro non sono sostenibili. La cessione del credito fiscale vede anche la centralità dello Stato nel contribuire fortemente agli investimenti, alleggerendo così il carico dei cittadini. Una misura come il superbonus, non basata sulla logica del debito, è di per sé restrittiva perché comporta il pagamento degli interessi. Sono questi alcuni degli esempi che portano a sostenere la validità della cessione del credito fiscale. Abbiamo poi il tema della sostenibilità nel tempo della misura del superbonus, che è un altro tema dibattuto. Vorrei ricordare ai colleghi del centrodestra, che forse non leggono le relazioni e non leggono le misure a supporto dell'introduzione del superbonus, la misura nata a maggio 2020 con il decreto-legge rilancio fu proposta per un tempo limitato (dicembre 2021) e con una copertura finanziaria fino a 34 miliardi di euro. poi state le proroghe successive, peraltro approvate da tutte le forze politiche, compresa Fratelli d'Italia, che ha sostenuto anche in campagna elettorale la proroga della

euro. Siamo stati tutti sostenitori e siamo tutti responsabili a questo punto di questa misura targata MoVimento 5 Stelle. Inoltre, l'errore metodologico che molti fanno, soprattutto del centrodestra, è l'inquadramento della misura. Infatti quando la misura è stata introdotta - io ero e sono fiero di essere stato partecipe di quel Governo di quel Governo e di aver sostenuto la cessione del credito fiscale - essa rientrava in una politica industriale che vedeva al centro il settore edile edile ed anche la valorizzazione centrale del patrimonio immobiliare. Con il settore edile e con la valorizzazione del patrimonio immobiliare del Paese noi abbiamo creato le condizioni per creare quel valore aggiunto su tutta la filiera del *made in Italy*. Abbiamo così fatto ripartire l'economia italiana, italiana, diventando anche il motore dell'economia europea, raggiungendo poi un PIL *record* in assoluto. assoluto. La sostenibilità del superbonus non deve limitarsi quindi solo a valutare gli aspetti contabili del dare, cioè la spesa sostenuta, ma deve andare a considerare un modello multidimensionale, che pone al centro della valutazione i costi insieme ai benefici. Quindi al dare della spesa vanno associati poi i benefici legati all'avere di quella spesa.

da istituti di ricerca, da associazioni, da ANCE, dai dottori commercialisti, dal Censis, da Nomisma, solo per citarne alcuni. Tra i benefici, troviamo un'alta capacità di investimento (la misura ha cubato 100 miliardi in tre anni; siamo fieri di questo); il suo prezioso contributo alla crescita *record* del PIL, pari a oltre il 12 per cento negli anni 2021-2022; oltre 100.000 nuove imprese nate e sorte solo nel settore dell'edilizia; un milione di posti di lavoro; 2 milioni di unità abitative coinvolte, considerando la media di appartamenti per condominio (altro che

secondo dati ANCE. Se però noi ascoltiamo l'Agenzia delle entrate, il gettito fiscale è stato notevolmente superiore, tanto che ANCE ha stimato un gettito fiscale pari al 74 Abbiamo poi l'emersione del lavoro nero, il risparmio energetico, il risparmio di interessi, la riattivazione del mercato immobiliare, il contributo alla realizzazione degli obiettivi della transizione *green* nel PNRR, la riduzione di CO2, i contenimenti

dove noi abbiamo da riqualificare circa cinque milioni di edifici. Vorrei ricordare che di di questi cinque milioni, un milione e mezzo di edifici sono stati costruiti prima del 1945 e ottocento addirittura prima del 1918. Come andremo a realizzare la riqualificazione di questi edifici? Con quali strumenti e con quali risorse andremo a recepire La direttiva case *green* è alle porte; noi adesso con questo decreto-legge cancelliamo tutto. Noi avremmo dovuto anticipare quelle misure necessarie per recepire la direttiva *green*. Ora il MoVimento 5 Stelle, ma - attenzione - anche la Lega e Forza Italia, che forse non dialogano tra loro e non dialogano con il Governo, hanno presentato dei disegni di legge, sia alla Camera che al Senato, cui affrontano il tema degli strumenti per realizzare la transizione *green* legata alle case. Sapete qual è l'assurdità? Tutte queste misure si basano sulla cessione del credito fiscale che oggi voi cancellate. (*(Applausi)*. Per tutte queste ragioni esprimo a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle la nostra contrarietà assoluta al provvedimento in discussione.

finalmente si torna alla normalità e a dare un quadro certo al settore, ma anche alle imprese e ai cittadini italiani e si fa un'uscita ordinata da strumenti straordinari. Non solo il 110 per cento, ma anche il bonus facciate, erano strumenti straordinari che, per onestà intellettuale, se fossero stati fatti bene, avrebbero avuto forse un senso in un periodo straordinario - grande crisi, Covid - ma - ahimè - non sono stati fatti bene. Non siamo più in un periodo straordinario: non c'è più *lockdown*, non c'è più la possibilità di fare sforamenti di bilancio infiniti, siamo tornati a fare bilanci normali. E come funziona il bilancio in un periodo normale? Beh, ce lo l'insegna qualcuno che di bilancio ne capisce: Luigi Einaudi, non so se qualcuno se lo ricorda. Nel 1919 Einaudi disse una cosa molto semplice: il Governo non ha un pozzo di San Patrizio. Il Governo non ha mica un pozzo di San Patrizio da cui cavare miracolosamente i mezzi onde colmare le perdite; non è che ci vuole uno scienziato. Mi perdoni, senatore Garavaglia, se la interrompo. Colleghi, vi sembrerà curioso, ma meno si è in Aula e più si sentono le voci di chi non sta intervenendo.

Allora che cosa non va? Abbiamo detto che queste misure avevano dei difetti. Che cosa non va in queste misure? Innanzitutto il costo abnorme: 140 miliardi - vedremo poi alla fine per un beneficio molto ridotto. Figuriamoci quante cose fai con 140 miliardi, è una cifra che si fa fatica a capire: con 4 miliardi fai una centrale nucleare, con 50 miliardi riempi tutti i Comuni di scuole nuove da 10-15 milioni l'una. È una cifra fuori da ogni misura. Inoltre, al di là del costo e del piccolo beneficio, è una misura super regressiva, perché ha beneficiato di questa misura soprattutto la fascia alta della popolazione, benestante, al Nord; quindi, mi stupisco che tanti non abbiano fatto anche questa piccola osservazione, visto che si parla tanto di riequilibrio Nord-Sud. soprattutto le seconde case e quindi, anche dal punto di vista ecologico, qualcuno mi deve spiegare qual è il beneficio di mettere il cappotto termico a una seconda casa al mare che si usa quindici giorni l'anno: zero, soldi buttati. Al netto di questo, poi ci sono le truffe. Le truffe, al di là della dimensione (vedremo poi fra qualche anno quante sono le truffe), hanno due dimensioni. La prima riguarda l'esistenza o no del credito fiscale sottostante, ceduto. I fondi stanno verificando titolo per titolo se esiste o no il lavoro dietro il credito fiscale. Se non c'è il lavoro, quel credito è un titolo tossico. Ci vorranno anni a fare questo lavoro.

con il trapano a girare l'Italia a vedere se c'è o non c'è il cappotto termico dichiarato e passeranno anni prima che si finirà di scoprire truffe, ma non è finita. Ogni tanto sentiamo parlare di condono e qualcuno se ne lamenta: ma cosa saranno mai quei 22 miliardi che nei prossimi anni non vengono incassati dallo Stato, se non un condono?

perciò è un'illusione credere che si possa avere qualcosa al di sotto del costo, cioè *gratis*. Tutto Tutto ciò che si può ottenere è pagare la differenza in un'altra maniera, il che è infantile, sempre citando Einaudi. Il problema però, oltre alle minori entrate, è il *deficit*. Sappiamo che lo Stato si finanzia con le entrate delle imposte e facendo debito, perché non basta quello che incassa per coprire la spesa: ogni anno facciamo *deficit*. Tre volte lo Stato non ha fatto *deficit*, due volte a fine '800, con la destra storica di Minghetti e Quintino Sella, e una volta nel 1925, con De Stefano. Tutte le altre volte lo Stato ha fatto *deficit.*

perfetto. In conclusione, sempre citando il nostro ottimo Einaudi, una misura così regressiva, fortunatamente finita, deve anche tener conto di un principio cardine, che dovrebbe interessare tutti noi, perché i Parlamenti nascono per decidere come si usano i soldi dei cittadini (nascono per questo, i Parlamenti). Piccolo concetto del 22 luglio 1919, sempre di Luigi Einaudi: lo Stato siamo noi; troppo spesso ci dimentichiamo che lo Stato siamo noi e che il Governo, in realtà, è un insieme di persone nominate da noi con certi incarichi. Non chiediamo dunque allo Stato e al Governo cose assurde: adesso cerchiamo di chiedere invece solo ciò che è capace di fare e avremo provveduto meglio ai nostri interessi. Ebbene, chiudendo questa misura misura straordinaria, fatta in modo sbagliato, stiamo facendo gli interessi nostri, quindi degli italiani.

a sostegno di un voto favorevole della Lega al decreto-legge in esame. Mi domando e domando ai colleghi, ovviamente per suo tramite, come mai proprio poche settimane fa, quando in quest'Aula abbiamo discusso - anche se per poco - e abbiamo poi votato ed è stata approvata la legge di bilancio, il Governo e la maggioranza non abbiano colto l'occasione per costruire un'uscita graduale e ordinata, condivisa perlomeno all'interno della stessa maggioranza. Mi sembra infatti di ricordare che punti di vista diversi nelle stesse forze di maggioranza, anche in occasione della discussione della legge di bilancio, si siano manifestati proprio su questa misura. Andava probabilmente costruita un'uscita graduale da una misura che indubbiamente - questo non lo sosteniamo noi o i colleghi del MoVimento 5 Stelle, ma lo dicono i dati - ha dato un suo forte contributo in senso anticiclico nella ripresa post-Covid del Paese. Così come è indubbio il contributo economico, è anche indubbio che, cambiata la fase - oggi per fortuna il momento emergenziale ce lo siamo lasciato quella misura avesse bisogno di un significativo tagliando, proprio per adeguarla ad un contesto e ad una contingenza che è diversa. Non è un caso infatti che molti dei nostri emendamenti alla legge di bilancio, che poi abbiamo riproposto nella discussione odierna in Aula, andassero proprio in questa direzione: costruire le condizioni per uscire gradualmente o modificare la misura Questa operazione, questa idea non l'abbiamo avuta soltanto noi; ho già ricordato come anche emendamenti di maggioranza in una direzione analoga siano stati presentati alla legge di bilancio, peraltro coerentemente con le promesse elettorali dei partiti che oggi sono al Governo; promesse elettorali che, come è stato sottolineato, sono state ampiamente tradite, sicuramente su questo punto. La maggioranza, per ordine del Governo, ha evidentemente bloccato, anche nelle settimane precedenti a quella odierna, il tentativo di diversi parlamentari di mettere ordine sulle scadenze, assicurando all'Aula della Camera e del Senato che il Governo sarebbe intervenuto con una misura più complessiva, con un decreto *ad hoc*. È stata questa la ragione per cui è stata messa la museruola anche ai parlamentari di maggioranza, facendo ritirare o bocciando tutti gli emendamenti che cercavano una via d'uscita più ordinata. Poi il provvedimento *ad hoc* complessivo è arrivato, è approdato oggi in Aula. Per generosità possiamo definire risibile. È stato approvato alla Camera senza modifiche rispetto al testo che il Governo ha licenziato in Consiglio dei ministri ed è arrivato in Senato con la stessa indicazione: vietato emendare, vietato proporre migliorie, vietato fare proposte, insomma, vietato ai parlamentari di opposizione e anche a quelli di maggioranza di fare il lavoro per cui siamo stati eletti dai cittadini. È lo stesso identico metodo con cui avete ignorato solo poche settimane fa, quando abbiamo discusso la legge di bilancio, le nostre proposte in materia di Irpef agricola ed oggi siete costretti a rimediare in fretta e furia sull'onda delle proteste con misure insufficienti ed estemporanee che immagino approderanno tra qualche settimana in quest'Aula. Sarebbe bastato, anche soltanto in piccola parte, accogliere le proposte e le preoccupazioni, come è stato già richiamato, delle associazioni di impresa e dei sindacati di settore. Solo qualche settimana fa, l'ANCE, Confedilizia e altre organizzazioni del settore che sono state audite in Commissione finanze alla Camera, hanno descritto la portata numerica, la dimensione del problema che ci troviamo di fronte. Solo parlando di condomini sono circa 40.000 i cantieri incompiuti, il 15 per cento del totale che è stato ammesso al 110. Ciò vuol dire 350.000 famiglie coinvolte, che oggi si trovano in difficoltà, per un valore di circa dieci miliardi. Il decreto che oggi ci avete presentato e che abbiamo discusso, a fronte di questi numeri, riesce a mettere insieme e a proporre uno stanziamento e un fondo di sedici milioni di euro. Praticamente, facendo due calcoli, si tratta dello 0,16 per cento del fabbisogno, ponendo peraltro un limite di reddito ISEE di 15.000 euro. ovviamente risibile, perché sfido qualunque collega a sostenere che famiglie con un ISEE di 20.000 o 30.000 euro, che hanno avuto accesso a questa misura, non siano famiglie in difficoltà. Non soddisfatti di questa barriera di reddito ISEE, il decreto insiste su un punto dal mio punto di vista ancora più odioso; restringe, cioè, le maglie agli interventi per l'abbattimento delle delle barriere architettoniche. Il decreto restringe di molto la possibilità di usufruire dei benefici per chi, ad esempio, abbia valutato in passato di apportare migliorie, con nuove tecnologie, rispetto a procedure per sollevare persone disabili da un piano all'altro. Questa restrizione sul tema delle barriere architettoniche suona alquanto cinica e beffarda, soprattutto in un momento momento in cui anche le forze di maggioranza insistono molto sul tema e sulla questione della disabilità. A me, sinceramente, tali restrizioni sembrano incomprensibili e ciniche. Noi abbiamo proposto diversi emendamenti, riproponendo delle priorità e dei ragionamenti, che abbiamo provato a suggerire anche durante la legge di bilancio. Anche per un'esigenza di natura conoscitiva, infatti, ogni legge del nostro Parlamento dovrebbe essere accompagnata da un sistema di valutazione dell'impatto, anche per lasciare al legislatore che verrà dopo di noi elementi di conoscenza su cui basare le proprie decisioni, che non siano soltanto una presunzione di efficacia o di inefficacia. Con emendamenti e con ordini del giorno abbiamo chiesto ad enti pubblici, ma indipendenti nella loro natura, come Enea, di quantificare, non solo per il passato, ma anche per il futuro l'impatto, non soltanto di natura economica, ma anche di efficienza energetica. fatto che gli emendamenti siano stati bocciati, ma mi risulta incomprensibile come mai anche impegni di natura più tenue, come ordini del giorno che avevano solo lo scopo di offrire elementi di maggiore conoscenza e consapevolezza, consapevolezza, non siano stati proprio presi in considerazione da questa maggioranza e dal Governo. mi avvio a concludere su un altro punto che ci sta particolarmente a cuore e che peraltro è stato oggetto di emendamenti presentati anche da altre forze di opposizione. individuare delle misure *ad hoc* e delle scadenze posticipate per alcune situazioni di grave difficoltà oggettiva, derivante da eventi come l'alluvione in Emilia-Romagna. Vi sono contesti territoriali che hanno sofferto, non per loro volontà o per la natura del provvedimento, ma per eventi avversi ed imprevedibili, conseguenze peggiori di altri. Procrastinare le scadenze, almeno per quei territori, sarebbe stato un segno di sensibilità e vicinanza a chi ha sofferto quelle situazioni che ci saremmo aspettati dal *premier* Meloni, che in prima persona si era detta disponibile realizzare cose che poi non abbiamo visto. Mi sembra che questi argomenti, queste motivazioni, siano più che sufficienti per giustificare il voto contrario del Gruppo Partito Democratico che si esprimerà, appunto, votando in senso contrario su questo provvedimento.

finalmente stiamo mettendo un punto ad una delle misure più disastrose degli ultimi decenni. *(Applausi)*. Anzi, purtroppo si tratta solo di un punto e virgola; gli effetti di questo catastrofico provvedimento graveranno infatti sulle casse pubbliche e sulle spalle dei cittadini ancora per molto tempo, grazie alle scellerate scelte di alcuni pessimi Governi passati. Questi governanti sono colpevoli di aver deliberatamente illuso, raggirato, ingannato il popolo italiano. *(Applausi)*. Un po' come la storia di Pinocchio: un gatto e una volpe o meglio, nel nostro caso, un comico e un avvocato. Gli hanno detto che lavorare non sarebbe servito, perché tanto i soldi nelle tasche sarebbero arrivati comunque, forse grazie all'albero degli zecchini d'oro. Affacciati da un balcone, lo hanno convinto che bisognava festeggiare, perché la povertà - pensate un po' - era stata abolita per legge. E soprattutto gli hanno raccontato che si sarebbe potuto procedere alla ristrutturazione della propria abitazione gratuitamente, come se le finanze statali venissero periodicamente rimpolpate da una sorta di manna dal cielo e non dipendessero invece dalle imposte pagate dagli onesti contribuenti. In altre parole, al motto «è gratis» qualche Governo passato ha ammorbato il mondo del lavoro, trasferendo un concetto pericolosissimo di un assistenzialismo diffuso, senza categorie di merito e di necessità, ed in pari tempo ha drogato il mercato sano dello sviluppo edilizio. Questo i dati lo dicono chiaro e forte. Da quanto emerso dalla relazione dell'Agenzia delle entrate, infatti, si evidenzia un impatto altamente negativo sui conti pubblici e sull'economia italiana, in quanto da marzo a settembre 2023 sono emersi altri 35 miliardi di crediti ceduti o scontati in fattura, che non erano previsti nei tendenziali di spesa. Oltre quattro miliardi di questi crediti, poi, si sono manifestati fasulli, con la conseguenza, tra le prime, che la scellerata iniziativa, alla data del settembre 2023, aveva già eroso i fondi della manovra finanziaria. Sono numeri che ho ricavato dalla relazione del professor Ruffini, fonte autorevole, che allo stato attuale non siete ancora riusciti a smentire. Continuo con questa triste giaculatoria. Il *bonus* per i lavori sulle facciate al 90 per cento doveva costare 5,9 miliardi, ma sta constando 26 volte e mezza di più. Per il superbonus 110 per cento si prevedeva una spesa di 35 miliardi, ma siamo quasi a 100. Tutti soldi che pesano sui conti del 2024 e per gli anni a venire. La piena dei vecchi bonus viene scaricata nella piattaforma dell'Agenzia delle entrate, tuttora fuori controllo; e potrebbero arrivare altre ondate nei prossimi mesi. A fine luglio 2023 mancavano ancora 20.000 condomini da finire, con lavori per 20 miliardi. Altre perdite miliardarie derivano dai crediti in circolazione che non troveranno un acquirente o che, per incapienza, non potranno essere scontati dalle imposte di chi li detiene, mettendo in conto anche le inevitabili crisi delle aziende e dei loro lavoratori. Potrei continuare all'infinito, ma mi rendo conto che sarebbe un accanimento anche nei confronti di chi all'epoca, dai banchi della minoranza, aveva segnalato queste anomalie e aveva cercato invano di far ragionare coloro che, incuranti del dopo, marciavano trionfanti verso il viale del baratro. Non azzardo un paragone iperbolico se definisco dunque il superbonus lo *tsunami* dell'economia, un ciclone che ha inciso negativamente in ogni settore, non solo edilizio; ha drogato il mercato, ha elevato i costi dei materiali, ha consentito a tutti indistintamente, anche ai proprietari delle seconde case di lusso, di godere di benefici correlati. Una frana che si è abbattuta. Questo commento non tradisce una malcelata soddisfazione per l'insuccesso dell'iniziativa, ma realizza invece la consapevolezza che governare significa innanzitutto decidere per il bene della collettività prendere decisioni talvolta anche impopolari *(Applausi)*, che chi è chiamato ad amministrare deve assumere senza essere influenzato dalle sirene del consenso spicciolo. È stato perpetrato consapevolmente un cortocircuito perfetto: la crescita abnorme di crediti legati ai *bonus* edilizi, oltre a rappresentare un grosso problema di bilancio - con la nuova classificazione Eurostat tutta la spesa si scarica sul primo anno e non può essere più spalmata come prima - ha anche congestionato le procure, che devono vagliare il profluvio profluvio di denunce per truffe derivanti dal distorto uso della misura. Non voglio entrare nelle dinamiche dell'autorità inquirente, ma è difficile stabilire il perimetro della violazione laddove mancano le regole, i decreti attuativi e i prezziari cambiano di continuo. Ebbene, anche questa volta il Governo Meloni, conti alla mano, si trova dunque a porre rimedio ai danni creati dai suoi predecessori, a dover governare pensando agli italiani del presente, ma soprattutto a quelli del futuro, figli e nipoti che a causa dei Governi precedenti nascono già pesantemente indebitati. *(Applausi)*. Il Governo Meloni ha l'ingrato compito del fanciullo che, nella favola di Andersen, svela la nudità dell'imperatore e ha l'altrettanto ingrato compito di gestire un Paese con la zavorra iniziale. Il Governo Meloni sceglie di mettere la parola fine ad alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia e alle continue circolari mensili, che dovrebbero essere esplicative, ma di fatto sono palesemente arzigogolate, incomprensibili e generatrici di nuove e più oscure circolari. Mettiamo consapevolmente la parola fine, cercando di salvaguardare le famiglie, le imprese che hanno confidato nella misura e avrebbero voluto farne un uso proprio. Per questo all'articolo 1 è stato previsto che le detrazioni rientranti negli interventi della disciplina del superbonus, sulla base degli stati di avanzamento lavori, per chi ha scelto lo sconto in fattura o la cessione del credito, non sono oggetto di recupero, in caso di mancata ultimazione dell'intervento.

che prevede l'istituzione di un fondo specifico, ma che non lasciava alternative. Di ciò ringrazio, a nome di Fratelli d'Italia, il Governo. Ancora una volta (l'ennesima), abbiamo dimostrato coerenza con le idee e con i principi che ispirano la nostra azione politica. Noi stiamo dalla parte di chi, anche nelle retrovie, certifica quotidianamente il proprio impegno per il Paese, non di coloro che, di fronte alle difficoltà collettive, intravedono l'occasione per un proprio tornaconto personale. Presidente, sono consapevole della lunga memoria di quest'Assemblea, ma non vorrei che prevalesse il ricordo selettivo. Ci tengo, quindi, a sottolineare che il Governo giallorosso ha favorito, con la manovra, la ristrutturazione di sei castelli e - si dice - di una fortezza. Aggiungo il commento degli illustri statisti che avevano sostenuto che l'incentivo fiscale sarebbe stato foriero del 40 per cento della crescita cumulata del PIL italiano nel biennio 2021-2022, poi dimostrato di superare l'1 per cento. Sarebbe fin troppo semplice smentire l'affermazione citando i dati dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha calcolato che il moltiplicatore del superbonus è di poco inferiore all'unità e che solo la metà dell'incremento è ascrivibile all'incentivo fiscale. Il tutto evidenzia un danno al Paese, che non ha portato una crescita economica, ma che è stato un fuoco di paglia, già esaurito con il tempo.

attorno al 20 per cento del totale dei crediti del *bonus*, e di restituire così giustizia ai cittadini e alle aziende oneste, i veri onesti, non quelli che si sono riempiti la bocca della parola «onestà» e hanno poi consentito questo intollerabile scempio della finanza pubblica.

Oscar Wilde diceva che i buoni propositi sono assegni che le persone firmano quando non c'è un conto su cui fare affidamento; aggiungo io che i cattivi propositi dei Governi che hanno impunemente licenziato i *bonus* edilizi sono cambiali in bianco che le generazioni future dovranno scontare.

nel modo meno rumoroso possibile. Senatore Sensi, attendiamo un attimo.

Signor Presidente, poche ore fa, ufficialmente per un arresto cardiaco, è morto Ihar Lednik, prigioniero politico in Bielorussia, in carcere da due anni per avere - così recita la sentenza contro di lui deliberatamente screditato con false informazioni e degradato l'onore e la dignità del dittatore Lukashenko in un articolo di giornale. Come se fosse possibile l'onore e la dignità di un dittatore. Si tratta del quinto prigioniero politico che muore dietro le sbarre del carcere bielorusso, dopo Vitold Ashurak (un altro arresto cardiaco), Mikalai Klimovich, Ales Pushkin, Vadzim Khrasko (morto appena un mese fa). Giornalista, sindacalista, componente del partito socialdemocratico bielorusso, Lednik era stato condannato a tre anni di colonia penale, dove è rimasto nonostante le sue condizioni di salute fossero più che precarie. Era un uomo mite e determinato, un giunco, ma di acciaio. Non so se sia un caso che le luci più abbaglianti della resistenza contro il regime di Putin

politica italiana, almeno per qualche istante, si è ritrovata ieri sera insieme - chi più e chi meno, ma insieme - in Campidoglio, non solo per ricordare, ma per dire il nome di Navalny, per farlo suonare come un talismano, uno scudo, come una fiammella di democrazia e libertà, *contra spem*, contro il realismo della fatica e il cinismo dell'indifferenza e dell'ignavia. Ne sanno qualcosa gli ucraini in trincea che combattono per la nostra vita. In questi Paesi di asfissia dei diritti civili e umani, perfino la forma più elementare della testimonianza, deporre un fiore, costa il carcere, la tortura, la pelle. Le piazze russe e bielorusse non si gonfiano più di protesta. La resistenza è esistenza; esistenza in vita fatta di gesti semplici, umani, gentili, e per questo eversivi, come vestire un colore o sopravvivere in una cella. Ad Alexei Navalny e Ihar Lednik va oggi dunque la nostra premura. Nelle carceri dove il regime ha sepolto i loro corpi esausti oggi continuano ad ardere della loro battaglia Vladimir Kara-Murza e Ilya Yashin. In Bielorussia sono oggi 1.422 i detenuti politici, attivisti, giornalisti.

Diciamoli i loro nomi. In queste ore, signor Presidente, sono dieci anni dalla rivoluzione ucraina della Euromaidan. Fu speranza e repressione, prologo in cielo, fragole e sangue di quello che stiamo vivendo come europei, di fronte sempre allo stesso nemico; dico nemico, non avversario. Un fiore per Navalny, un fiore per Lednik, dunque, Presidente: la vostra esistenza ha fatto frutto, la vostra resistenza continua. Senatore Sensi, io credo che quest'Aula sia uno dei luoghi più adatti per ricordare a tutti i doveri i doveri sulla libertà di opinione e di espressione e il dovere di tutti noi di esserci. La ringrazio anche per aver ricordato che tutte le forze politiche sono intervenute

Presidente, voglio fare ancora una volta in quest'Aula un appello per Julian Assange da dodici anni rinchiuso ingiustamente. Queste ore sono drammaticamente importanti per il suo destino. In questi giorni terminerà l'udienza e l'Alta corte di giustizia britannica dovrà decidere sul ricorso sul ricorso presentato contro l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. Julian Assange ha fatto il suo lavoro, rivelando crimini di guerra e aprendo gli occhi a tante persone sull'orrore delle guerre in Iraq e in Afghanistan. Quello che è successo lo ha poi portato ad essere detenuto in un carcere di massima sicurezza e, se verrà estradato, passerà probabilmente il resto della sua vita, avendo una condanna di centosettantacinque anni, prigioniero degli Stati Uniti.

se Julian Assange vivrà o morirà, ma soprattutto se vivrà o morirà l'informazione libera e indipendente. Rilevare crimini non è un crimine. Per questo continuiamo a dire libertà per Julian Assange.